L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.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

in tempi molto stretti. Abbiamo provato a fare del nostro meglio e credo di poter dire che, grazie anche al supporto prezioso e sempre puntuale e preciso dei nostri Uffici, abbiamo svolto un buon lavoro. Lo abbiamo fatto in una dialettica, naturale per quanto accesa, tra maggioranza e forze di opposizione dato dal Parlamento, seppure in tempi contingentati, sia stato decisamente in grado di migliorare il provvedimento.

abbiamo fatto inserendo norme importanti e soprattutto - come dirò in seguito nella relazione - modificando il provvedimento che il Governo poi ha inserito, con un emendamento, all'interno del decreto-legge n. 221. Lo abbiamo fatto a seguito anche di una presa di posizione della Commissione, con una lettera

il Parlamento riesca a dare il proprio contributo. Ovviamente la mia relazione si soffermerà soprattutto sul contributo dato dalla Commissione nel modificare e migliorare il provvedimento. Quindi proverò, per quanto sia noiosa come relazione, a dire, articolo per articolo, dove siamo intervenuti e come abbiamo migliorato il provvedimento. 1 reca l'ulteriore proroga al 31 marzo 2022 dello stato di emergenza nazionale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da Covid-19. prevede che il capo dipartimento della Protezione civile e il commissario straordinario per l'emergenza adottino anche ordinanze finalizzate alla programmazione della prosecuzione in via ordinaria delle attività necessarie al contrasto e al contenimento dell'epidemia in corso. Durante l'esame in Commissione è stato presentato un emendamento da parte del Governo, contenente, oltre al decreto-legge

Il nuovo articolo 2 novellando l'articolo 1 del decreto-legge n. 33, sopprime l'obbligo di quarantena precauzionale prevista in via generale in caso di contatto stretto con un soggetto positivo al virus e prevede in sostituzione, laddove resti la negatività al virus, un regime di autosorveglianza e l'obbligo di indossare dispositivi FFP2 e FFP3. L'articolo 3-*bis*, novellando l'articolo 9 del decreto-legge n. 52, introduce la definizione delle certificazioni verdi cosiddette *green pass* base e *green pass* rafforzato, rispetto alle quali vengono conformate le modificazioni contenute nei due decreti-legge nn. 221 e 229. L'articolo 4 reintroduce l'obbligo dal 25 dicembre 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge, fino al 31 gennaio 2022, anche in zona bianca e anche nei luoghi all'aperto di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e, fino al termine dell'emergenza, l'obbligo di mascherine FFP2 per gli spettacoli e per gli eventi sportivi. All'articolo 4-*bis* si impegna il commissario straordinario a definire, consultate le associazioni dei produttori di dispositivi di sicurezza, e di intesa con il Ministero della salute, un protocollo con le farmacie e altri rivenditori autorizzati per assicurare, fino al 31 marzo 2022, la vendita a prezzi contenuti dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2. In Commissione sono state inserite due novità: la deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie anche per le strutture sanitarie interessate direttamente o indirettamente nell'emergenza da Covid-19 e l'istituzione di un tavolo tecnico presso il MISE per la pianificazione, anche in futuro, degli approvvigionamenti dei dispositivi di protezione. Gli articoli 5 e seguenti, così come modificati dall'emendamento governativo, prevedono un'elencazione delle attività soggette a obbligo di certificazione verde di tipo base rafforzato, che vengono così presentate in forma più chiara e trasparente per i cittadini. In particolare si prevedono, fino al 31 marzo (termine di cessazione dello stato di emergenza), anche i corsi di formazione privati svolti in presenza tra le fattispecie il cui accesso è subordinato al possesso di un certificato verde di tipo base. L'articolo 5-*bis* reca, fino alla cessazione dello stato di emergenza, un ampliamento delle fattispecie di ambiti e attività il cui accesso è riservato ai soggetti in possesso di un certificato verde Covid-19 generato esclusivamente da vaccinazione o da guarigione. Resta ferma la possibilità di svolgimento e di fruizione senza il possesso di un certificato verde per i minori di età inferiore a dodici anni e per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione. un emendamento in Commissione è stata poi estesa la capienza per eventi sportivi fino al 75 per cento all'aperto e al 60 per cento al chiuso. All'articolo 5-*ter* viene prorogata fino al 31 marzo 2022 la validità delle disposizioni che disciplinano l'obbligo di possesso ed esibizione delle certificazioni verdi Covid-19 cosiddette base in ambito scolastico, educativo e formativo, nonché nell'ambito della formazione superiore. L'articolo 5-*quater* prevede l'obbligo del possesso del cosiddetto super *green pass* a decorrere dal 10 gennaio 2022 per l'accesso e l'utilizzo di mezzi di trasporto. L'articolo 5-*quinquies* opera una proroga al 31 marzo 2022 dell'applicazione delle norme transitorie che richiedono il possesso di un certificato verde Covid-19 ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, sia nel settore pubblico che in quello privato. prevede la proroga delle norme transitorie in materia di certificati verdi per l'accesso agli uffici giudiziari dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari e dei componenti delle commissioni tributarie. L'articolo 6 vieta, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge fino al 31 gennaio 2022, gli eventi e le feste che implicano assembramenti in spazi all'aperto. Per il medesimo periodo sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. L'articolo 7 disciplina l'accesso dei visitatori alle strutture residenziali socio-assistenziali, socio-sanitarie e *hospice* per il periodo compreso tra il 30 dicembre 2021 e il 31 marzo 2022. L'articolo 9 proroga al 31 marzo 2022 la somministrazione a prezzi contenuti di *test* antigenici rapidi. L'articolo 10 modifica la disciplina della piattaforma informativa nazionale istituita per le attività di vaccinazione contro il Covid-19. L'articolo 11 definisce una misura urgente per il controllo dei viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2. L'articolo 12 proroga fino al 31 dicembre 2022 l'applicazione della normativa già vigente per il 2021, che consente la somministrazione nelle farmacie aperte al pubblico, da parte dei farmacisti, dei prodotti vaccinali contro il Covid, con relativa definizione grazie a tutti

conservazione delle dosi vaccinali per esigenze nazionali. L'articolo 15 apporta alcune modifiche alla disciplina relativa all'applicazione Immuni. L'articolo 16 proroga fino al 31 marzo 2022 i termini delle disposizioni legislative di cui all'allegato *a)* del decreto-legge in esame. In Commissione è stato esteso al 31 marzo 2022 il divieto di applicare ai gestori dei servizi di trasporto pubblico sanzioni o penali a causa delle minori risorse o minori percorrenze effettuate. Viene poi esteso al 2022 lo scomputo delle spese per i contratti a tempo determinato della Polizia negli enti locali delle limitazioni finanziarie in materia di pubblico impiego. Viene inoltre prorogata al 15 giugno 2022 l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relativa all'anno accademico 2020-2021. Infine, l'articolo 17 reca una disciplina transitoria per lo svolgimento di lavoro agile da parte dei cosiddetti lavoratori fragili nei primi due mesi del 2022. A questo proposito, in Commissione è stata estesa al 31 marzo 2022 l'equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva per i lavoratori fragili. Mi sia consentita una considerazione finale prima di concludere. Ovviamente - è inutile dirlo - il provvedimento in esame viene convertito in un tempo diverso

Credo che, rispetto a questo, sia nostro dovere mantenere alta l'attenzione. Ritengo anche che, ancora una volta, nelle circostanze date e sicuramente in tempi non facili per la politica, per stare ai tempi con un'epidemia che cambia in maniera veramente repentina, abbiamo fatto il miglior lavoro possibile nelle condizioni date.

Se la legge - e segnatamente l'articolo 24 del codice della Protezione civile - prevede che lo stato di emergenza debba avere una durata massima di dodici mesi (prorogabili,

mesi. Lo stato di emergenza - lo dice la parola stessa - ha un senso per fronteggiare situazioni imprevedibili ed eccezionali. Con il decreto-legge che oggi siamo chiamati a convertire il Governo, dopo una serie innumerevole di provvedimenti analoghi, ha in realtà normalizzato l'emergenza. l'emergenza. Lo stato di emergenza è, però, una misura estremamente grave che comprime

Proprio perché si tratta di principi costituzionali, questi possono ragionevolmente essere compressi soltanto in un giudizio di comparazione di fronte - appunto a situazioni eccezionali. Purtroppo la pandemia si è protratta per tanti mesi anche a causa dell'incapacità del Governo di fronteggiarla con misure adeguate,

che pure noi di Fratelli d'Italia abbiamo chiesto continuamente, inascoltati: mettere in sicurezza i trasporti; rendere obbligatoria la mascherina FFP2 nei luoghi affollati, nei mezzi di trasporto, nelle metropolitane, e soprattutto sui treni regionali; la ventilazione nelle scuole. Per mesi lo abbiamo chiesto e soltanto nell'ultimo periodo, finalmente, avete cominciato a darci ragione,

come sappiamo - ormai in quest'Aula la voce dell'unica opposizione è considerata un fastidio, e credo che lo stiano dimostrando tutti i colleghi dall'estrema sinistra fino alla destra: siamo un fastidio chiedo scusa se continuiamo a ostinarci a credere nella democrazia; chiedo scusa se ci ostiniamo a credere che questa Assemblea dovrebbe essere un luogo di confronto anche fra opinioni diverse, ma questo è

continuare ad affastellare norme su norme sempre più confuse, sempre più contraddittorie, sempre più complicate? Ci vorrà un manuale di cento pagine ormai per ogni cittadino per sapere come può andare a fare la spesa; come può andare al cinema o a teatro; viaggiare sui mezzi di trasporto ed esercitare le minime libertà costituzionali che pure gli dovrebbero essere sempre garantite.

che lavora all'aperto o per un'impresa familiare dove ci sono solo genitori e figli e non estranei, è una delle norme assolutamente irragionevoli;

Questo vuol dire che forse avevamo ragione noi, ascoltando quegli esperti che ci dicevano che il vaccino non impedisce la circolazione del virus, che si può contagiare ed essere contagiati anche se si ha la terza dose e - come dimostra, purtroppo, la situazione drammatica di Israele - anche se si ha la quarta dose.

di uccidere, per il terzo anno consecutivo, uno dei principali fattori di sviluppo e di prodotto interno lordo, che è il turismo italiano.

Qui non si tratta più di ragionare in modo pragmatico su ciò che è utile e su ciò che non lo è. Non si tratta più di fare un bilanciamento tra i diversi interessi che pure sono in campo, perché c'è certamente l'interesse per la salute - siamo i primi a dire che la salute va assolutamente tutelata - ma c'è anche l'interesse per l'economia. Oggi tutto il mondo sta cercando di uscire da questo dilemma per garantire quella ripresa economica di cui c'è assolutamente bisogno. E, invece, voi continuate con questa religione per cui non è più possibile discutere nel merito. Cara Presidente, mi lasci concludere con una considerazione: è veramente scandaloso che nella discussione di questi giorni siano entrati anche i figli, o meglio le figlie, di due *leader* politici, Giorgia Meloni e Matteo Salvini. I sacerdoti della religione del politicamente corretto non si vergognano nemmeno di trascinare nella polemica politica una scelta individuale di genitori che, insieme ai medici e ai pediatri, sono liberi di scegliere senza diventare oggetto di dibattito politico o peggio. E mi riferisco anche ai colleghi del PD, come il senatore Marcucci, che si dovrebbe vergognare... Senatore Balboni, si rivolga sempre alla Presidenza e non direttamente al fatta anche da oltre i due terzi di tutti i genitori italiani. Ecco le ragioni per cui chiediamo di non passare

che possono dirsi di opposizione. Si tratta quindi di una propaganda che svia l'attenzione dei cittadini che ci seguono.

è qualcosa che non ha eguali - l'abbiamo detto più volte su questo tema - nella storia repubblicana. Le caratteristiche di uno stato di emergenza sono sicuramente la gravità e l'eccezionalità; se poi l'eccezionalità diventa ordinaria amministrazione, allora siamo di fronte a qualcos'altro, visto che abbiamo compresso in maniera incredibile le libertà personali e abbiamo stravolto la vita delle persone, delle famiglie e delle imprese. Serve dunque la responsabilità, la responsabilità, che ci porta qui oggi a votare a favore, e che ci ha portato ieri in Commissione a presentare un ordine del giorno che la Lega ha fortemente voluto, a prima firma del collega Augussori, ordine del giorno con cui si chiede al Governo l'impegno di rivedere, con equilibrio, ragionevolezza e proporzionalità, le norme che ci siamo e abbiamo imposto agli italiani. I dati vanno in una precisa direzione grazie alla responsabilità di chi non ha contrapposto semplicemente un chiudiamo tutto a un apriamo tutto, ma ha lottato - come ha fatto la Lega - per la singola norma, per la singola categoria, per la singola iniziativa. Ogni giorno ogni attività un po' più aperta o meno chiusa cambia la vita delle persone. Abbiamo dunque voluto ieri un ordine del giorno e abbiamo presentato degli emendamenti - alcuni sono stati accolti - che vanno in questa direzione, perché anche un giorno può fare la differenza nell'allentare non solo semplici misure, ma un vero e proprio cappio che sta al collo, spesso anche sul lato economico, di tantissime attività. Un'altra parola che va aggiunta è «tempestività»: questo va fatto subito va fatto subito e, quindi, chiediamo non solo quotidianamente di poter rivedere le misure, ma di farlo anche oggi in Aula. Faccio l'esempio concreto di un emendamento che è stato bocciato ieri in Commissione, ma che come Lega abbiamo scelto di ripresentare, che riguarda alcune delle manifestazioni a cui tutti siamo più legati e che da Nord a Sud accomunano il nostro Paese. In esso si chiedeva, su sollecitazione dei sindaci, di poter allentare le misure in zona bianca per consentire manifestazioni come la processione

per dette manifestazioni in zona bianca significa andare in una direzione di riapertura e ripartenza del nostro Paese. Il Governo ha dato parere contrario, l'emendamento è stato bocciato e l'abbiamo ripresentato in Aula. Allora, chiederei al Governo di

il proprio parere, anche ai colleghi della Toscana, della Sicilia, della Sardegna e di tutte le Regioni dove si svolgono manifestazioni come quelle enunciate, che per centinaia di anni hanno rappresentato la nostra tradizione - rinunciare alla tradizione è il primo passo per rinunciare a se stessi e alla propria storia

Diamo un segnale e facciamolo partendo dalla nostra tradizione e dalla nostra essenza. Se non lo dovesse fare il Governo, mi auguro che possa rivendicarlo e farlo il Parlamento.

ieri mi è stato segnalato come anche in Senato sia stato approvato un provvedimento che fa seguito al *super green pass* e che introduce le stesse regole che valgono per i luoghi di lavoro: alcuni parlamentari, non vaccinati, si troveranno dunque nella condizione di non poter partecipare ai lavori dell'Aula e di non poter svolgere la funzione per cui sono stati votati da centinaia di migliaia di persone. In questo modo si priva il Paese di una parte della sua rappresentanza, fatta di persone che sono sane - ripeto, sane - e che con un semplice tampone potrebbero verificare la propria contagiosità; limitazione che non viene fatta a chi si è vaccinato, sebbene è evidentemente dimostrato che il vaccino non elimina la contagiosità. credo che tutti voi ricorderete i falsi proclami sulla validità del vaccino e sulla sua efficacia contro la trasmissività del virus. Credo inoltre che sia palese a tutti come parificare il nostro compito a quello di tanti altri lavoratori significhi sminuire l'alto ruolo che ci è stato assegnato. Non credo che si debba evidenziare con superbia il ruolo che ricopriamo, ma almeno riconoscere l'alto compito che c'è stato assegnato e che cerchiamo di svolgere nel modo migliore. Ricordo a tutti che pochi giorni fa, durante l'elezione del Presidente della Repubblica, è stata creata una postazione esterna che ha permesso anche a chi aveva il Covid, come il sottoscritto, Mi rammarico che lo stesso trattamento non sia stato riservato alle persone sane e in particolare alla deputata Cunial, che invece ha commesso il grave peccato di non essere vaccinata, come se i diritti costituzionali dipendessero dall'essere vaccinati. I diritti costituzionali - non dobbiamo mai dimenticarlo - sono diritti propri di tutti i cittadini e privare un rappresentante del popolo del suo diritto di rappresentanza credo sia un fatto gravissimo, cui non avrei voluto assistere. Ma le assurdità non finiscono qui. Oggigiorno uno straniero che giunge in Italia può accedere a ristoranti e mezzi di trasporto avendo fatto un semplice tampone e, dunque, non essendo necessariamente vaccinato. Con un semplice tampone uno straniero potrà viaggiare sui nostri treni, mentre un non vaccinato italiano non potrà farlo, come se gli italiani fossero cittadini di serie B. Questa semplificazione per gli stranieri, pur nella sua assurdità e discriminazione, non riuscirà ad ogni modo a compensare le immani perdite del settore turistico, terrorizzato da regole draconiane e in continuo cambiamento, che hanno orientato i turisti che amavano il Bel Paese verso altri lidi e, in particolare, dove quelle misure non sono state adottate. Basta poco per trovarli, perché *super green pass* e obbligo vaccinale siamo stati quasi i soli a introdurli in tutta Europa. Quasi ovunque anche le misure più lievi del *super green pass* sono state eliminate, anche in Paesi dove il contagio ha mietuto numerose vittime. Quasi ovunque si riconosce la minore pericolosità della variante Omicron, che è quella ampiamente dominante nel nostro Paese. Mi stupisco come si continui a sostenere la validità del *super green pass* e dell'obbligo

È mia opinione che la cosa migliore sarebbe oggi far decadere il decreto-legge e riconoscere con onestà che le misure che abbiamo preso non sono state efficaci o lo sono state in misura molto ridotta. Una cosa, però, è certa e ce lo ha segnalato Amnesty International, l'associazione che da decenni si batte per i diritti umani in tutto il pianeta. Amnesty, il 19 gennaio, sollecita il Governo ad ancorare i propri interventi ai principi di legalità, legittimità, necessità, proporzionalità e non discriminazione. Qualsiasi politica di salute pubblica, inoltre, deve essere basata sull'evidenza scientifica più aggiornata e verificabile, motivata da comprovate ragioni oggettive e accompagnata da metodi di comunicazione chiari e trasparenti. Sembra dunque evidente che da Amnesty alcuni interventi adottati dal nostro Paese non solo sono stati giudicati illegali, illegittimi, non necessari, non proporzionali, ma anche discriminanti. La politica di salute pubblica è inoltre parsa non basata sulle evidenze scientifiche più aggiornate e verificabili e non accompagnata da metodi di comunicazione trasparenti. È facile verificare la ragione di queste critiche: ancora oggi riceviamo giornalmente un bollettino dei decessi, ma non sappiamo se si tratti di persone morte per Covid-19 o con Covid-19, tutte messe nello stesso calderone. Sappiamo poco dei decessi e delle reazioni avverse legate alle vaccinazioni, che purtroppo ci sono e sono stati minimizzati. Tuttavia, anche in questi giorni si legge che gli aspetti positivi della vaccinazione sono maggiori di quelli negativi, cosa che posso anche condividere. Ma non vorrei che qualcuno di voi si trovasse nella condizione di dover rincuorare una famiglia che ha perso un familiare, magari una bambina, o ha una bambina, o ha subito reazioni avverse permanenti. E le miocarditi sembrano molto più frequenti di quanto dichiarato. Abbiamo continuato a ripetere fino alla nausea che il vaccino era sicuro, benché sia ancora in fase sperimentale e non sappiamo se potrà generare reazioni avverse a lungo termine. continuo ad avere impressa l'immagine dell'amministratore delegato della Pfizer che dice che le prime due dosi di vaccino non hanno quasi effetto e che l'efficacia di un certo rilievo con la terza dose. È noto, però, che il vaccino è stato creato per la variante Delta e lo stesso amministratore delegato ribadisce che un vaccino specifico per la variante Omicron sarà pronto in marzo. Qualsiasi persona con un minimo di cervello si rende, però, conto che vaccinare a marzo, quando i contagi sono in forte calo, e fare un richiamo a luglio-agosto, quando i contagi sono quasi assenti, è un controsenso sanitario. Ovviamente, non è un controsenso l'interesse economico per le ditte farmaceutiche, che hanno guadagnato e continuano a guadagnare miliardi con i vaccini. probabilmente, si sarà sviluppata una nuova variante, dato che la pandemia non si ferma vaccinando il 100 per cento dei cittadini di un Paese: cosa impossibile, che non è riuscita ad alcun Paese. Ci sarà sempre una parte della popolazione che, per i più svariati motivi, non vorrà vaccinarsi e noi tutti dobbiamo rispettare quella volontà, anche se si tratta di singole persone. È assurdo introdurre introdurre l'obbligo vaccinale e contemporaneamente chiedere alle persone di firmare una liberatoria in caso di reazioni avverse come avviene ora. Purtroppo, con il *super* *green pass* abbiamo negato,

dove sono conservati i propri risparmi, misura che colpisce ovviamente le persone anziane, che non hanno dimestichezza con l'accesso telematico. La cosa più grave, comunque, è stato impedire alle persone di poter svolgere il proprio lavoro, impedendo persino l'accesso ai mezzi pubblici. Il lavoro è un diritto fondamentale e mi chiedo come tutti voi possiate sostenere una misura volta a compiere un vero e proprio ricatto verso una fascia, seppur ridotta, della popolazione. Noi tutti dovremmo lavorare per il rispetto dei diritti fondamentali di ogni persona e non mi risulta che il diritto al lavoro e all'accesso al posto di lavoro abbia cessato di essere un diritto fondamentale del nostro Paese,

tematiche, ma cercherò di condensare in pochi minuti alcuni concetti che sono emersi non soltanto dalla discussione del presente provvedimento in Commissione, ma anche dal cosiddetto affastellamento normativo che le Aule del Parlamento vedono, avendo al proprio esame provvedimenti relativi alla gestione dell'emergenza pandemica. Noi veniamo, con questo provvedimento, a gestire ancora lo stato d'emergenza e, conseguentemente, gli strumenti che sono ad esso collegati: quindi, il *green pass* e il regime delle vaccinazioni. l'azione di Governo si sia dovuta confrontare con una situazione grave. E, nonostante i numeri siano oggi positivi, nel senso che pare che la curva sia effettivamente in decremento e andiamo verso una risoluzione di quelle che sono

nei confronti dei nostri cittadini, che molto spesso non comprendono la bontà delle norme che andiamo ad approvare, quando esse ovviamente sono buone. Cito l'esempio di una cittadina

semplicemente perché l'amministrazione comunale cui si rivolgeva non ha voluto nemmeno visionare la documentazione di esenzione vaccinale.

ma perché non ci si è arrivati prima? Questa è quanto il nostro Gruppo, i nostri parlamentari, cercano di portare all'attenzione del Governo; un'attenzione che bisogna prestare nei momenti in cui si propongono degli emendamenti, che non sono di parte o semplicemente finalizzati ad acquisire consenso elettorale, come magari altri possono pensare.

identità, perché qualcuno, all'interno della compagine governativa, evidentemente non ha voluto prestare adeguata attenzione. *(Applausi)*. Noi siamo consapevoli, perché siamo convintamente al Governo, che però questa attenzione tornerà ad esserci e che quindi anche questo tipo di problemi potranno essere risolti. Auspichiamo altresì che possano essere risolte alcune distorsioni, quali ad esempio quelle all'interno del mondo dello sport.

cosa che mi sta particolarmente a cuore - la possibilità di far praticare sport anche ai minori di anni dodici che si sono vaccinati, quindi che hanno scelto di vaccinarsi, che però nei quindici

le nostre riunioni che lo sport fa bene, che aiuta la salute e ci accompagna verso una ripresa non soltanto psicologica, ma anche fisica, perché non dare la possibilità anche a questi ragazzi di esercitare legittimamente e nel pieno delle loro capacità lo sport inteso come promozione personale, sociale e sportiva? Queste sono le attenzioni che chiediamo al Governo. Queste sono le attenzioni

sicuramente e pienamente il loro stato di cittadini. È un richiamo che faccio al Governo, lo faccio personalmente e credo che lo si possa fare come Aula parlamentare. Chiedo davvero che questa attenzione venga portata dal Sottosegretario ai Ministeri competenti e in particolare al ministro Speranza affinché possa capire che certe proposte non sono propagandistiche e politiche, ma semplicemente proposte di buonsenso.

stiamo esaminando l'ennesimo decreto-legge che si occupa della situazione sanitaria che vive il nostro Paese. Dobbiamo dire però qualcosa di importante che non deve passare inosservato. Stiamo convertendo un decreto-legge del 24 dicembre 2021 e, nelle more, il Governo, valutata la curva epidemiologica, ha ritenuto di intervenire per mitigare quelle che nel momento della sua adozione sembravano misure necessarie e che invece la curva epidemiologica rassicurante ha dimostrato poter essere attenuate. È così, non può essere diversamente. L'andamento della curva epidemiologica mette nelle condizioni il Governo, d'intesa con il Comitato tecnico scientifico, di apportare quelle modifiche che rendano più sopportabili

che la vaccinazione rende immune il soggetto, nella maniera più assoluta. Sicuramente è stato detto e accertato che la vaccinazione limita di molto le conseguenze dannose dell'epidemia;

proroga lo stato di emergenza, che ci auguriamo il 31 marzo possa terminare, ma anche i poteri del capo della Protezione civile e della struttura commissariale, però apporta delle modifiche significative. Per esempio, per i titolari di *green pass* che vengono in contatto con positivi non è più necessaria la quarantena, ma l'utilizzo per dieci giorni della mascherina FFP2, quindi un autocontrollo del soggetto. Sono state modificate alcune situazioni all'interno della scuola, che credo sia stata la struttura più penalizzata: i nostri ragazzi purtroppo pagheranno nel tempo le conseguenze che questa epidemia ha riversato sulla scuola,

durante il giuramento del Presidente della Repubblica, per una maggiore considerazione del Parlamento e un maggiore coordinamento con il Governo. all'esame parlamentare all'ultimo momento diventa difficile poter dare un contributo sostanziale. Noi, per esempio, abbiamo modificato come meglio abbiamo ritenuto il presente decreto-legge, ma i colleghi della Camera probabilmente dovranno approvarlo così come il Senato lo

prevedeva la possibilità, per il commissario straordinario, di chiamare al tavolo della crisi i produttori

che il commissario straordinario chiami in una concertazione i produttori italiani di mascherine e che nel tavolo tecnico istituito possano essere rappresentate un elemento da chiarire: la collega Pirovano aveva presentato un emendamento di buon senso, che prevedeva la necessità di mitigare i prezzi delle mascherine per i bambini. Anche su questo il il Governo ha espresso un parere contrario a nostro avviso non fondato, anche se lo abbiamo rispettato. Anche in questo caso, nelle audizioni che abbiamo tenuto in 1a Commissione i produttori italiani di mascherine hanno detto di essere in grado di avviare una produzione di mascherine per bambini e di impegnarsi a mitigarne il prezzo. Mentre oggi basta entrare in una qualunque farmacia o parafarmacia per vedere messaggi pubblicitari che parlano di mascherine per bambini (che pare non esistano, però così viene scritto), che vengono vendute a un prezzo non mitigato; questo reca sicuramente un danno. È importante anche un emendamento approvato a favore dei lavoratori fragili. fragili. Questo, per esempio, è un caso in cui c'è stato un eccellente coordinamento tra il Parlamento, il Governo e i Ministeri: poiché mancavano i fondi per coprire questa esigenza, è venuto il Ministero del lavoro e si è fatto carico totalmente delle somme necessarie.

a quella europea, è cresciuta in maniera maggiore; e questo un significato ce lo deve pure avere. Questo sicuramente è il frutto dei tanti sacrifici che hanno fatto i nostri imprenditori, i nostri lavoratori e i nostri concittadini; dobbiamo anche prenderci i meriti e non soltanto farci carico delle situazioni negative che abbiamo dovuto sopportare. provvedimento necessario e utile, che si può migliorare. Abbiamo avuto l'impegno da parte del vice ministro Sileri, che ha partecipato a parte dei lavori, di

di vaccinazione. E ce ne sono tante altre, come il trasferimento dalle isole al continente. Sono ancora in cantiere tante altre iniziative, che il Governo si è impegnato ad approfondire e a inserire nei prossimi provvedimenti. Quindi, il nostro non può che essere un giudizio positivo su questo provvedimento, nell'auspicio che in seguito si possano migliorare e limitare al massimo o eliminare completamente le restrizioni e i sacrifici che i nostri concittadini hanno dovuto fare nel nostro

siamo in discussione generale sul provvedimento in esame, relativo alla proroga dello stato di emergenza e alle misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia. In merito vorrei proporre alcune riflessioni e soprattutto far emergere delle criticità non tanto inerenti alle misure previste, ma soprattutto nel metodo. Questo anche grazie alla presenza del Sottosegretario, che magari può riferire al Governo. Partiamo dalla considerazione principale, cioè che la salute è il bene primario di ognuno di noi e che il ruolo di chi governa è fare di tutto per preservarla, che è giusto e doveroso avvalersi di persone competenti in campo medico e scientifico, per fare in modo che le decisioni prese abbiano una base scientifica e soprattutto riescano a mitigare i rischi. Ma poi le decisioni politiche di fatto sono di competenza del Governo o, più precisamente, del Ministero della salute. Non voglio contestare le misure adottate, perché, se di fatto almeno quest'inverno non siamo stati costretti a *lockdown*, vuol dire che hanno avuto efficacia; e questo è un dato positivo, anche per quanto riguarda le vaccinazioni. L'appunto che voglio fare è sul metodo. Comprendo che la situazione non sia facile e che le decisioni non vengano prese a cuor leggero; ma per prendere queste decisioni ci siamo avvalsi di esperti, che, con i loro studi, possono prevedere

Credo che determinate affermazioni fossero supportate dai dati di virologi o scienziati. Quindi di fatto, all'inizio dell'autunno, si potevano ipotizzare le misure da mettere in campo, come le chiusure di determinati esercizi, e quindi anche prevedere di supportarli nell'immediato con efficaci ristori. Cioè la politica: io ti chiudo, io ti pago.

ma anticipare l'intenzione avrebbe forse evitato a questi esercenti la programmazione di eventi, l'acquisto delle merci, la preparazione dei locali e le pratiche necessarie per effettuare gli eventi (che sono tutti costi).

il decreto, e vedremo quando le risorse saranno erogate ai beneficiari che, nel frattempo, dovranno trovare le risorse per pagare le fatture. Un'altra criticità emersa dai decreti riguarda la decisione di abbassare la validità del *green pass* da nove a sei mesi. Anche questa decisione ha influito negativamente sul mondo del turismo, già in difficoltà in questo periodo. Come ho più volte ribadito, il turismo è fatto di programmazione e flussi turistici che determinano il buon andamento della stagione. Questa scelta ha di fatto messo in difficoltà il turismo invernale, già logorato dal *lockdown* dello scorso anno. Infatti, il turismo invernale nel periodo delle settimane bianche è per lo più sostenuto dal turismo estero, pari a circa l'80 La decisione di diversificare la durata del *green pass* rispetto agli altri Stati europei ha avuto come conseguenza una marea di disdette, obbligando alcuni alberghi a chiudere

caso, però, mi preme ringraziare il ministro Garavaglia, che si è subito attivato per trovare una soluzione a questa problematica che permetterà di salvare il resto della stagione.

che stanno dando il massimo per garantire le cure a tutti i cittadini. Sono convinta che bisogna trovare delle soluzioni che consentano alle strutture sanitarie di non andare in criticità. Sappiamo quante persone attendono interventi urgenti, che purtroppo sono stati

oggi all'esame dell'Assemblea, pubblicato il 24 dicembre 2021, nella relazione esplicitava l'intento di recare disposizioni necessarie a fronteggiare con immediatezza l'evolversi della situazione epidemiologica nell'attuale contesto di rischio, che impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario ed urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività. Infatti, in tale data l'ondata di contagi dovuta alla variante omicron iniziava la sua impennata anche in Italia, con una decina di giorni di ritardo rispetto alla situazione che già si delineava in altri Paesi europei come la Gran Bretagna, la Spagna, la Danimarca e altri.

l'emergenza connessa all'evolversi della situazione epidemiologica, integrando ulteriormente il quadro delle misure delineato dal decreto-legge del 24 dicembre. Come primo nuovo provvedimento, si prevede il prolungamento dello stato di emergenza nazionale per ulteriori due mesi, dal 31 gennaio fino al 31 marzo. Tale previsione va in controtendenza rispetto a quanto operato dagli altri Paesi europei: uno stato di emergenza che si protrae oltre i due anni per fronteggiare una pandemia che certo non si preoccupa di rispettare i confini nazionali dovrebbe essere parimenti adottato anche dagli altri Paesi europei; invece, vediamo altri Paesi a noi vicini come la Spagna eliminare lo stato di emergenza precedentemente adottato, altri Paesi come la Gran Bretagna o la Svizzera non hanno mai adottato lo stato di emergenza, la Danimarca lo ha abrogato da cinque mesi. Se ne potrebbe dedurre che lo stato d'emergenza in Italia viene mantenuto per coprire altre inefficienze del Governo. Si prolunga lo stato di emergenza perché il sistema sanitario è ancora in affanno. Significa che le misure e gli interventi finora adottati non sono adeguati e sufficienti ad assicurare alla popolazione un sistema sanitario efficace per tutelare la salute dei cittadini.

un elevato livello di vaccinazione; secondo il «Financial Times», che mantiene una classifica aggiornata sulla base dei dati forniti dai siti governativi dei diversi Paesi, l'Italia è al secondo posto in Europa, seconda solo alla Danimarca, per dosi di vaccino somministrate. L'Italia ha vaccinato in percentuale più del Portogallo, più del Belgio, più della Francia, più della Germania, più dell'Austria, più della Spagna, più della Gran Bretagna (e potrei continuare elencando tutti i Paesi europei), ha vaccinato molte più persone in percentuale rispetto ad Israele, molte di più rispetto alla Svizzera. Anche per quanto riguarda la distribuzione della terza dose, l'Italia è in testa alle classifiche, avendo già raggiunto il 60 per cento della popolazione. La Gran Bretagna ha raggiunto il 56 per cento, la Germania il 55 e la Francia con la terza dose è arrivata al 50 Per quale motivo, allora, visto il successo della campagna vaccinale, l'Italia continua a performare peggio per quanto riguarda il contrasto alla pandemia? L'Italia, con i suoi attuali 360 decessi in media al giorno, ossia 6,15 decessi per milione di popolazione contro i 4,19 della Francia, i 3,12 della Gran Bretagna, l'1,64 della Svizzera, l'1,38 della Germania, manifesta la situazione peggiore in Europa per decessi. A fronte del più alto tasso di vaccinazione, ha ancora il più alto tasso di mortalità per Covid-19 in Europa. Mi domando e domando al Governo, quali sono le nuove ulteriori misure, in aggiunta alla campagna di vaccinazione, che si intendono intraprendere per ridurre il tasso di mortalità per Covid-19. Questo prolungamento dello stato di emergenza quali obiettivi si propone di raggiungere per risolvere definitivamente questa situazione critica di alta letalità, al fine di tutelare meglio la nostra popolazione? Tornando al provvedimento in esame, all'articolo 3 e con il successivo emendamento governativo il Governo si preoccupa di modificare la durata della validità delle certificazioni verdi Covid-19 a far data dal 1° febbraio 2022. Mi domando: come può essere volta a fronteggiare con immediatezza l'evolversi della situazione epidemiologica una misura che entra in vigore quaranta giorni dopo la pubblicazione? Dove sta l'immediatezza dell'azione di contrasto? La previsione di modifica si spiega nella relazione - è volta a consentire la somministrazione della terza dose anche a coloro che, *medio tempore*, non l'hanno ancora ricevuta, e nel contempo a evitare l'inefficacia delle certificazioni verdi Covid che risulterebbero scadute con l'entrata in vigore della nuova normativa. Si tratta di una normativa esclusivamente burocratica: non è chiaro cosa impedisse ai cittadini di ottenere la terza dose e cosa con questa norma sarebbe stato facilitato. Piuttosto, i cittadini a quel tempo richiedevano in massa la terza dose, mentre le somministrazioni non erano disponibili e venivano calendarizzate con difficoltà. Secondo un modo elementare di ragionare si penserebbe che, a fronte di un'emergenza sanitaria per la quale ancora è necessario un contrasto e un'azione governativa importante, vengano poste in essere misure che mettano in campo maggiori risorse per quanto riguarda la cura e la prevenzione. invece il decreto-legge in esame si preoccupa fondamentalmente di mettere pesanti restrizioni alle libertà personali a quella piccola fascia di cittadini che consapevolmente e lecitamente ha deciso di non avvalersi della vaccinazione.

dai 30 ai 39 anni e dai 40 ai 49 anni sono le fasce di popolazione per le quali il virus, a parte le situazioni di fragilità personale, è stato affrontato dai sistemi immunitari personali degli organismi umani in modo molto efficace, pertanto l'incidenza della letalità e di patogenicità grave sono state bassissime, anche nel periodo di assenza dei vaccini. Invece, il decreto-legge introduce previsioni di accanimento proprio per queste fasce di popolazione giovanile che costituiscono oltre il 70 per cento delle persone che oggi risultano ancora non vaccinate. Viene vietato il consumo di cibi e bevande al banco al chiuso e nei servizi di ristorazione, l'accesso agli alberghi e alle altre strutture ricettive, agli spettacoli aperti al pubblico, a eventi e competizioni sportive; viene proibito l'accesso ai musei e ai luoghi della cultura, alle piscine, ai centri natatori, alle palestre e ai centri sportivi, ai centri benessere, alle feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, ai corsi di formazione privati, se svolti in presenza. Non è proprio facile capire dove sta il buon senso nell'applicare queste restrizioni molto dure, uniche in Europa, che ci posizionano al livello più alto al mondo per *stringency index*. Oltre alle limitazioni sulla libertà personale, tali limitazioni per combattere la pandemia hanno portato al crollo di attività in bar, ristoranti, pizzerie, agriturismi, cosa che ha travolto conseguentemente interi settori dell'agroalimentare e *made in Italy*. Coldiretti stima in 5 miliardi di euro l'ammontare di cibi e vini invenduti, e nel 2022 il *trend* è in peggioramento. Secondo Epat Ascom Torino, bar e ristoranti a Torino

l'incomprensibile dissonanza delle norme attualmente in vigore. Con l'obbligo della certificazione verde o *green pass* per musei e monumenti nei luoghi del turismo e della cultura non si può più entrare. Presidente, le chiedo per favore ulteriori trenta secondi per poter terminare. Nel nostro Paese, l'accesso alla cultura dovrebbe essere sempre incentivato e non ostacolato. Un gruppo di 20 scuole di danza si è riunito chiedendo alle istituzioni politiche di fare un passo indietro sulla normativa legata al *green pass*, perché il disagio dei giovani e delle ragazze sta aumentando e non si può andare avanti in questo modo. Perfino le squadre di calcio *under* 17 chiudono. Un uomo trentottenne si è dato fuoco in piazza a Oderzo perché non possedeva il *green pass* ed era stato multato. Chiedo al Governo di retrocedere rispetto a questa applicazione abnorme del *green pass* rafforzato, perché è evidente che non è una misura sanitaria e va a comprimere le libertà in modo violento sulle persone non soggette particolarmente alla patologia Covid-19, e rischia di aggravare danni dal punto di vista economico e anche della tenuta psicologica di bambini e nelle fasce

Signor Presidente, approfitto, apparentemente fuori tema, per esternare la mia amarezza per aver perso l'occasione, prima in legge di bilancio e adesso in sede di conversione del provvedimento unificato con l'emendamento del Governo per non aver saputo prenderci cura di chi si è preso cura, riconoscendo almeno un ristoro alle famiglie dei medici che, soprattutto durante la prima parte della pandemia, quando mancava di tutto (dal piano pandemico ai dispositivi di protezione individuale) e poco si sapeva di come affrontare il virus, con spirito di abnegazione hanno cercato di limitare, talvolta anche a scapito della loro stessa vita, gli effetti pandemici per i loro pazienti.

per ragioni ignote sia stato declassato a non prioritario, mentre a suo tempo, tanto per fare un esempio, sono stati trovati i fondi per i rifugi che salvano gli animali selvatici, molto meritoria ma dal mio punto di vista di priorità molto successiva a quella del ristoro di coloro che hanno salvato vite umane. Abbiamo perso due battaglie, ma non possiamo permetterci di perdere la guerra, pur nella consapevolezza che nulla potrà restituire all'affetto delle loro famiglie coloro che hanno perso la vita. Ma in loro memoria non tralasceremo nulla, anzi cercheremo di riproporlo in ogni dove, passando dalle parole ai fatti, ben prima del 18 marzo,

talvolta la classe medica è sottostimata rispetto a quanto effettivamente fa per il bene comune Entrando nella prospettiva evolutiva del provvedimento in discussione, ci insegna che dobbiamo essere lungimiranti, perché gli imprevisti, soprattutto nel campo sanitario, sono una variabile da tenere in considerazione ancora più che in altri settori. E non possiamo più permetterci di rincorrere la realtà, dovendo approcciare con metodo la prevenzione e il recupero dei ritardi nelle cure, a onor del vero già intollerabili ben prima della pandemia, in un in un quadro di visione sistemica, di prevenzione proattiva e di governo dei rischi individuali e collettivi, perché altrimenti ci troveremo di fronte ad un'ecatombe annunciata, con disposizioni incisive per rendere effettiva l'analisi predittiva e i sistemi di sorveglianza indicati, ma tuttora inattuati. occorre agire efficacemente con meccanismi molto persuasivi sul monitoraggio delle risorse, sui controlli e sulla responsabilità dell'intera filiera,

ci fa ritenere che la nostra fiducia al Governo, sebbene con qualche criticità di percorso e pur se si è andati un po' lunghi, era ed è ben riposta. Non deludeteci con il ristoro dei medici, diamo un senso anche alle parole del Presidente. È una prospettiva decisamente sfidante in termini di revisione ordinamentale, a garanzia dell'effettiva attuazione della missione 6 del PNRR, con un innovativo governo della sanità e nuove regole di ingaggio degli erogatori, compresi i medici di medicina generale, anche per ciò che riguarda l'integrazione proattiva fra medicina ospedaliera e territoriale, andando a ridurre l'incidenza dei rischi di patologie, non solo infettive, con una rete accreditata e a contratto di continuità assistenziale per livelli di intensità e tempestività di cura: su questo, nonostante gli apprezzabili sforzi, dovrebbe incidere un po' più marcatamente in valutazione e controlli di appropriatezza e sicurezza, in una cornice di piena responsabilità istituzionale. Lo stesso dovrebbe valere anche per l'adesione consapevole alla profilassi vaccinale, perché l'accresciuta fiducia dei cittadini nello Stato dovrebbe indirettamente superare molte delle perplessità sulla sicurezza e l'efficacia dei vaccini; come non smetterò mai di sottolineare, noi siamo tra coloro che ritengono che bisogna convincere per non costringere e uno degli argomenti più forti per convincere chi esita ed è contrario al vaccino è che lo Stato si assuma fino in fondo la responsabilità degli eventuali effetti avversi. *(Applausi)*. Dal nostro punto di vista un grande passo in avanti è stato fatto, anche per quanto riguarda l'impatto applicativo delle misure previste dal decreto-legge in conversione, con l'articolo 20 del decreto sostegni-*ter*, posto che si è finalmente palesato il concetto che non si può imporre un obbligo, nemmeno in forma surrettizia, senza assumersi le responsabilità delle eventuali conseguenze: dal 27 gennaio, grazie alla spinta della Lega, tutto questo è norma. Agire in prevenzione e promozione della salute della persona, della famiglia e della collettività attraverso l'adesione consapevole è dunque un'altra battaglia che dobbiamo saper combattere e vincere tutti insieme ne va del nostro futuro -, coniugando tutela della salute e libertà fondamentali secondo etica e responsabilità.

approfitto della discussione generale su questo provvedimento di proroga dello stato di emergenza - e speriamo di poter dare per scontato che sia l'ultima, per motivi sia di ordine giuridico che di ordine epidemiologico per lasciare a verbale alcune brevi considerazioni. La pandemia volge al termine, ovunque in Europa si abbandonano le misure restrittive prese o non si prendono le misure restrittive annunciate. La stessa relatrice ha sottolineato che il decreto-legge ma dovrei dire i decreti-legge, visto che il decreto-legge n. 229 del 2021 è confluito come emendamento nel n. 221, di cui trattasi - è ormai sorpassato dagli eventi. Ovunque in Europa ci si conforma alle sagge parole attribuite a Keynes: «Quando i fatti cambiano, cambio le mie opinioni. Lei cosa farebbe?». parole che, però, Keynes non ha mai detto (le ha dette Samuelson), ma che hanno un senso di per sé. Perdonatemi la sottolineatura sulla paternità della citazione, che non è solo un eccesso di feticismo erudito, ma è anche un modo per entrare nel vivo di un tema che sento di dovere e so di poter portare alla vostra attenzione: la preoccupante regressione culturale, che rischia di essere uno dei lasciti più pesanti e persistenti di questa pandemia; una regressione che ha preso le preoccupanti forme della compressione di ogni libero dibattito, in questa e in tutte le altre sedi, a beneficio di un ricorso totalizzante e totalitario al principio di autorità, all'*ipse dixit*. Quando quello che si dice diventa meno importante di chi lo dice, è facile che ci si avvii su strade senza uscita, soprattutto considerando che nel Medioevo *ipse* era Aristotele scientifico, nella qual cosa - mi perdonino tutti gli interessati - io non riesco a vedere un enorme progresso, se devo valutare il contributo di questo organismo alla luce degli strumenti che la mia formazione scientifica mi offre per giudicare i colleghi di disciplina non affine: la validità delle previsioni e la coerenza interna delle affermazioni. I giornalisti si sono divertiti - e io non voglio annoiarvi - con il repertorio di piroette e previsioni fallaci che questo organismo ci ha fornito. Torno sulla mia preoccupazione. Mi preoccupa l'analogia fra l'uso che una certa politica ha fatto della ha fatto della "scienza" e quello che da tempi risalenti sta facendo dell'Europa: l'Europa, prima, e la scienza, poi, sono diventati i mezzi attraverso i quali una classe politica si è sottratta alle proprie responsabilità, tra l'altro facendo di questi mezzi un uso sempre curiosamente asimmetrico. La scienza è stata utilizzata per chiudere, ma si recalcitra ad usarla per aprire; la scienza è stata utilizzata per imporre obblighi che si sono rivelati, poi, scientificamente infondati, ma ancora non se ne vuole prendere atto. Purtroppo - agganciandomi anche alle considerazioni della collega Cantù - il primo risultato dell'aver elevato ad alfa e omega del nostro dibattito, anche politico, questa paradossale fede nella scienza

Un'asimmetria analoga - sempre nel contesto del provvedimento che siamo analizzando - vale per la cosiddetta Europa, che poi, giova ricordarlo, sarebbe l'Unione europea. Il lasciapassare Covid-19 nasce con il regolamento UE 2021/953 come strumento per facilitare la libertà di movimento ed evitare odiose discriminazioni; è in quello spirito che personalmente espressi il mio voto favorevole in questa Aula il 16 giugno 2021: all'epoca sembrava necessario favorire la libera circolazione dei cittadini europei, per non uccidere la stagione turistica. L'applicazione che se n'è fatta, però, è andata in un'altra direzione e dobbiamo dircelo: lo strumento è stato utilizzato per limitare la circolazione dei cittadini italiani e ha dato adito a una serie di comportamenti odiosamente discriminatori e di continue intollerabili violazioni della *privacy*, anche di criminalizzazione di cittadini che stavano semplicemente esercitando un proprio diritto. Tra l'altro, ciò ha portato danni notevoli, che sono stati evocati in questa discussione generale, a numerose attività economiche. L'interrogazione del collega europarlamentare Antonio Rinaldi su come la Commissione intendesse intervenire per contrastare questi comportamenti discriminatori è rimasta inevasa. I regolamenti europei si applicano quando servono, per esempio come col *bail in*, ad azzerare risparmi dei cittadini italiani; si interpretano quando servono a difendere la loro libertà. Questa è una curiosa asimmetria. Dobbiamo riappropriarci, perché ne siamo capaci, della nostra capacità di giudicare i provvedimenti dai loro risultati. io devo dire che mi è molto difficile, anche in un'ottica comparativa internazionale, dare un giudizio positivo del *green pass* nella versione che abbiamo sperimentato in Italia, col suo corredo di obblighi, sulla cui dubbia legittimità costituzionale si diffonde autorevolmente il professor Alessandro Mangia in uno dei suoi ultimi interventi. Gli emendamenti, che la Lega ha presentato in questa sede e che presenterà in occasione delle prossime numerose scadenze di decreti affini, sono orientati a rendere meno vessatorio questo strumento. Ciò che però la Lega ha chiesto autorevolmente, per bocca dei suoi Capigruppo, è che esso venga definitivamente abbandonato con la fine dello stato di emergenza, perché ci preoccupa che la nostra vita sia affidata a un lasciapassare digitale in un Paese che non si è ancora posto il tema di recepire in Costituzione la tutela dell'identità digitale della persona, oggetto di un disegno di legge depositato dall'onorevole Morelli alla Camera. Un Paese in cui non si tutela nemmeno quel diritto minimo che è la capacità di effettuare e ricevere pagamenti elettronici e non si evita di condannare alla morte civile chi, per qualche motivo, si vede rifiutare l'apertura di un conto da un istituto bancario, come chiede da tempo il senatore Siri, con un disegno di legge di puro buon senso su cui ancora attendiamo il parere al Governo. In teoria, le parole d'ordine sono *digital* ed *inclusive*, ma poi, in pratica, l'intera infrastruttura digitale viene utilizzata per escludere e questo ci preoccupa. Ci preoccupa affidare la nostra esistenza o lasciapassare digitale in un Paese in cui non esistono presidi legislativi forti contro l'eventualità di vedere la propria identità digitale menomata o azzerata, ma anche in un Paese le cui infrastrutture informatiche hanno dimostrato di essere molto permeabili. Qui nel Lazio, sempre per restare in tema sanitario, se ne è avuta dimostrazione l'estate scorsa, col collasso, a causa di un attacco di *hacker*, dell'infrastruttura della sanità regionale, con tutti i problemi che poi ne sono conseguiti.

Se vogliamo recuperare competitività verso questo importante e, per certi versi, preoccupante concorrente, non dobbiamo inseguirlo sulla sua strada, quella del sistema dei crediti sociali, ma dobbiamo continuare ad affermare la nostra via verso il progresso, che è quella della tutela, sempre e in ogni sede, della libertà. La libertà, non la repressione, hanno garantito all'Europa la sua eccellenza e ha reso possibili le tante rivoluzioni scientifiche e tecnologiche che ci assicurano oggi livelli di benessere impensabili anche solo un secolo fa. Proseguiamo sulla strada della libertà. *(Applausi)*.

ed è fondamentale approcciarvisi con valutazioni attente e ponderate, considerato il quadro attuale, non solo dal punto di vista sanitario, ma anche economico e sociale. Va ricordato che quello che noi oggi chiamiamo *green pass*, come ha ricordato già il senatore Bagnai, è nato come strumento per agevolare il movimento transfrontaliero all'interno dell'Unione europea. Abbiamo poi deciso di estenderne l'utilizzo, attribuendogli la funzione di strumento di sanità pubblica. In questo momento, però, abbiamo il dovere di capire il fine dell'ampliamento del suo utilizzo in particolare e del suo mantenimento in generale. Ogni progetto necessita di un obiettivo. Dobbiamo, quindi, porci la domanda: qual è l'obiettivo che ci poniamo, nel breve e medio periodo, con un uso ancora più restrittivo di questa certificazione verde? A mio avviso, il rischio che corriamo, inasprendo ulteriormente le misure, è di minare la tenuta sociale del Paese, già fortemente provato dalla pandemia, unitamente ad una depressione della domanda interna, in un momento in cui, tra l'altro, i flussi di visitatori dall'estero sono fortemente ridotti. Girando per le nostre città, si osserva un Paese lacerato, depresso e purtroppo diviso. Tante misure legate al *green pass*, impattano soprattutto sui giovani, futuro del nostro Paese. Nei momenti difficili l'unità è un elemento fondamentale, che va perseguito con ogni mezzo. Questo è un elemento che non può non essere considerato. Non possiamo ignorare che l'estensione del *green pass* ha effetti importanti sulla contrazione della domanda interna, considerando che la spinta al consumo non è influenzata solo ed esclusivamente dalla disponibilità economica; un'atmosfera generale depressa e tesa influenzerà negativamente le scelte di consumo relative, ad esempio, allo svago. Il rafforzamento di una misura di natura emergenziale tende a generare stati di ansia nella popolazione con ricaduta proprio sui consumi. Come possiamo spiegare ristoranti vuoti con il 90 per cento di cittadini con il *super* *green pass*? A questo si aggiunge il tema dei turisti stranieri. Siamo certi che l'immagine che stiamo dando non sia quella di un Paese caratterizzato da innumerevoli restrizioni da evitare come luogo di vacanza? Anche perché questo avviene in un momento in cui Paesi vicini si apprestano ad eliminare o comunque ridurre fortemente l'impiego del *green pass*. più che mai dobbiamo essere consapevoli che parlare di spesa per le vacanze e il tempo libero non è essere frivoli o mancare di rispetto ai deceduti bensì porre attenzione a settori fondamentali dell'economia reale. Dietro ad ogni rinuncia a spendere sul nostro territorio ci sono famiglie che si impoveriscono, bambini che non avranno un'alimentazione adeguata, ragazzi costretti a interrompere gli studi, procrastinazione di scelte familiari che, prima o poi, impatteranno pesantemente sul nostro sistema Paese. Quello su cui dobbiamo concentrarci in questo momento è dare un segnale di ripartenza vera che non aggiunga limitazioni e complicazioni per chi lavora e favorisca la circolazione monetaria. È importante che ci impegniamo quindi a trovare soluzioni stabili che non puntano semplicemente a mettere delle toppe, bensì a creare le condizioni per una ripresa economica duratura. La contrazione della domanda interna a causa dell'ondata della variante Omicron, avviene in un momento in cui tra l'altro sono state introdotte forti limitazioni alla possibilità di cessione dei crediti con il decreto-legge sostegni-*ter* e antifrode. Cessione dei crediti significa sostegno alla circolazione di beni e servizi e quindi all'economia reale, obiettivo per cui mi sono impegnata nel corso del mio mandato, depositando due disegni di legge relativi alla cessione dei crediti fiscali e alla creazione di una piattaforma per lo scambio degli stessi, attualmente in esame nella Commissione competente. La gravità della situazione è tale che non può non essere affrontata se non con strumenti straordinari. Abbiamo bisogno di un'apertura mentale che introduca strumenti innovativi. Solo così saremo in grado di dare un messaggio forte di speranza ad una popolazione fortemente provata, incoraggiandola a credere nel futuro del nostro Paese. Non possiamo più trincerarci dietro misure palliative che già sappiamo non essere in grado di affrontare in modo risolutivo i problemi legati all'economia reale. Il superbonus 110 per cento è stato una palestra per sperimentare un modo nuovo di concepire il credito d'imposta, elevandolo a vero e proprio volano grazie a tutti chi con onestà si è approcciato al superbonus producendo effetti positivi sia sull'economia che sulla tutela ambientale in un momento particolarmente buio. Sarebbero proprio Sarebbero proprio questi ultimi a pagare il prezzo più alto di una limitazione allo strumento. Onorevoli colleghi, infine, nel ricordare a me stessa che dobbiamo agire in modo razionale e che la storia ci giudicherà per le scelte odierne, vi chiedo siamo certi di avere chiaro l'obiettivo che andiamo a perseguire con la conversione di questo decreto-legge e se siamo certi che stiamo perseguendo fini di tutela della sanità pubblica. E ancora: siamo sicuri che le regole che stiamo imponendo non stiano inducendo uno stato di stress tale nella popolazione che renderà difficile un ritorno alla normalità? Vi chiedo infine se siamo pronti ad affrontare i mesi che verranno con apertura mentale disancorandoci dagli schemi tradizionali, inidonei per fronteggiare la situazione economica attuale. attuale. Auspico, colleghi, in questo momento un dibattito sano, sereno e ponderato a tutela di tutta la popolazione italiana. Signor Presidente, mi unisco alle considerazioni svolte dalla collega Cantù riguardo alla vergognosa circostanza di non essere riusciti in tutto questo tempo a riconoscere un indennizzo minimo ai familiari dei medici e del personale medico in generale che ha perso la propria vita a causa della disorganizzazione, della disinformazione, della della mancanza di dispositivi sufficienti a proteggerli nella prima e anche nella seconda ondata di questa epidemia. Lo faccio dopo aver condiviso il provvedimento in Commissione e in tutte le successive occasioni in cui si è tentato di convincere il Governo a fare una cosa assolutamente normale, indispensabile, dignitosa. Devo anche dar ragione al collega Airola e non me ne vogliano gli altri. In effetti, ascoltando il dibattito, l'opposizione in quest'Aula Sottosegretario che rappresenta il Governo - va veramente molto oltre Fratelli d'Italia. L'opposizione verbale,

bisogna fare attenzione perché si scambia il verde con il rosso, insomma si scambia il voto a favore del Governo con quello contrario. *(Applausi)*. Senza scomodare Senza scomodare un grande siciliano come Sciascia, questa gente lui l'avrebbe chiamata "quaquaraquà", ponendoli cioè all'ultimo livello nella classifica degli uomini di quel grande uomo che era Sciascia. Do quindi ragione al collega Airola, perché in effetti Fratelli d'Italia è l'unico partito di opposizione che poi vota coerentemente con quello che dice. Questo è vero. Ci sono anche altri che fanno opposizione verbale e poi si allineano a quanto stabilisce il Governo.

e viene qui in Aula a prendersi tutte le giuste considerazioni fin qui ascoltate, c'è solo da esprimere umana considerazione, ci mancherebbe. Personalmente io non lo farei.

generale. Colleghi, oggi abbiamo di nuovo a che fare con provvedimenti che agiscono sul versante delle restrizioni e li andiamo a convertire in presenza di una realtà dell'epidemia che ci vede assolutamente soccombenti. Non è un'esagerazione verbale dire che continuate a emanare e a convertire provvedimenti mortiferi. Questo è un Governo che rispetto alla pandemia ha esercitato un'azione mortifera e non è un'esagerazione, perché in tutti i passaggi della pandemia, fin dall'inizio, l'Italia ha registrato e continua ancora oggi a registrare il record dei decessi.

e non si vergognano di farlo. Siamo davanti a una circostanza drammaticamente rilevante: abbiamo messo in ginocchio la nostra economia con risultati drammatici sul nostro prodotto interno lordo, abbiamo impedito l'esercizio di libertà fondamentali, abbiamo anche impedito la libertà di parola e di un confronto sereno e normale su temi essenziali, ottenendo come risultato il *record* dei morti, ancora oggi. E ancora oggi andiamo in televisione e veniamo in Parlamento a raccontare che dobbiamo continuare a fare le stesse cose fatte fino a oggi, che sono state mortifere. E di tutto questo non ci si vergogna, neanche davanti a se stessi, davanti allo specchio, davanti alla propria coscienza. coscienza. Rappresentante del Governo, le cose da cominciare a fare, perché le fanno anche gli altri, ottenendo risultati egregi, fare la ventilazione meccanica nelle aule, che costa quattro spicci e va fatta subito; potenziare i trasporti per evitare l'assembramento dei ragazzi (che non si proteggono con le mascherine, perché sono ragazzi) dentro gli autobus del trasporto scolastico; sviluppare le terapie domiciliari, perché è per questo motivo che abbiamo il *record* dei decessi. *(Applausi)*. La gente che non viene curata a casa,

dalla prima versione del virus, quando ormai il virus è totalmente mutato? Sottosegretario, non facciamo il tracciamento; e non fare il tracciamento significa perdere completamente il controllo della pandemia. Questo è il motivo per cui, tra gli altri, abbiamo il *record* dei decessi. Non facciamo neanche il sequenziamento, cioè non sappiamo oggi se una persona positiva al Covid, perché ha fatto un tampone (rapido o molecolare che sia), ha una variante Omicron o Delta o una nuova variante, perché è possibile che ci siano nuove varianti. Noi non sequenziamo e - attenzione - questo non lo dice il senatore Zaffini in Aula oggi,

Ancora oggi i medici di medicina generale non sono coinvolti e purtroppo ce ne sono tanti che raccontano stupidaggini. Non facciamo lo *screening* anticorpale, che altri Paesi fanno. Prima di procedere ad altre somministrazioni e di diventare

A che serve, quando da tutte le parti c'è scritto che gli anticorpi che derivano dalla malattia evidentemente sono ben superiori, migliori, performanti e immunizzanti degli anticorpi da vaccino (peraltro vaccino vecchio)? Perché abbiamo comprato dieci dosi di vaccino a testa in Europa? Il Governo questa cosa ce la può dire? Perché abbiamo comprato dieci dosi del vecchio vaccino? E perché continuiamo a somministrare il vecchio vaccino? È legittimo sospettare che dobbiamo semplicemente esaurire le scorte? È legittimo sospettarlo? Potrei parlare per un'altra mezz'ora e dire le cose che gli italiani tutti i giorni si chiedono. Presidente, la ringrazio del tempo che mi ha concesso, mentre qui lampeggia il microfono.

la fase critica della pandemia sembra volgere al termine. Ciò significa, però, non che sia finita l'emergenza, bensì che dobbiamo affrontare questa nuova fase con la massima cautela. Ce lo chiedono i cittadini i cittadini e le imprese che stanno vivendo una fase piuttosto interlocutoria, anche a causa dell'incerto quadro geopolitico internazionale all'interno del quale l'Italia sta necessariamente seguendo con grande preoccupazione la tensione gravissima tra Russia e Ucraina, che potrebbe davvero incidere in maniera devastante sulle nostre vite. L'Europa e l'Italia, in particolare, non possono permettersi di volgere lo sguardo altrove. L'approvvigionamento energetico, dal cui costo dipendono le vite delle imprese (in particolare, quelle medie e piccole) e - conseguentemente - la sopravvivenza delle famiglie ci deve far riflettere con attenzione. Il decreto-legge che ci accingiamo a convertire deve essere inteso in tutta la sua complessità. Lo abbiamo detto più volte: dalla pandemia non si esce da soli e non si esce se non considerando quelli che dovrebbero essere i valori fondanti di una società, ai quali si è peraltro richiamato anche il presidente Mattarella nel suo discorso di insediamento: solidarietà, diritto al lavoro e riduzione della diseguaglianza. In una parola: dignità dovuta a ogni essere umano. Il decreto sull'emergenza, dunque, riguarda tutti poiché definisce per l'ennesima volta quanto sia necessario dare per non mettere a repentaglio la salute di tutti a causa del richiamo di alcuni a quel valore sublime della libertà. il quale ci spiega quanto la libertà obblighi a prendere decisioni e le decisioni comportino dei rischi (nel nostro caso, il rischio di non tutelare abbastanza i più deboli, i più fragili e i più esposti in tutti i sensi). Il provvedimento disciplina con chiarezza l'accesso dei visitatori alle strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie e che comporta disagi importanti. Si tratta però di misure a nostro avviso necessarie per il contenimento della diffusione del virus in luoghi dove ci sono concittadini fragili a cui abbiamo il dovere di pensare. Le Istituzioni hanno il dovere di tutelare la salute di tutti, da cui dipende anche il nostro benessere. Quanto abbiamo acclamato - lo ha sottolineato anche il presidente Mattarella - un vaccino

Farci vaccinare è qualcosa che dobbiamo a chi non ce l'ha fatta, a quei più di 150.000 morti e a quegli operatori della sanità che hanno lavorato e continuano a lavorare con turni massacranti negli ospedali per curare anche coloro che, prima di ammalarsi di Covid anche in modo grave, schernivano noi vaccinati, permettendosi di dubitare della scienza e della ricerca. Con il provvedimento in esame è stato cercato un equilibrio tra tutte le forze politiche del nostro Emiciclo: un equilibrio faticoso, ma credo che possiamo ritenerci soddisfatti. Ringrazio tutti per l'approccio collaborativo e per aver contribuito a definire le regole che determinano questa nuova fase che abbiamo cominciato o stiamo per vivere. Ringrazio gli Uffici, che si sono spesi con generosità anche per sostenere il lavoro delle Commissioni. Spesso in quest'Aula c'è stato qualche richiamo ad altri Paesi. In questa fase in cui l'emergenza non può ancora dirsi del tutto superata, l'Italia ha saputo affrontare le difficoltà meglio di altri Paesi. Le regole severe hanno avuto la forza di prevenire il peggio: le chiusure di attività, già fortemente provate. Noi, a differenza che in altri Paesi, ci siamo presi la responsabilità di pensare ai cittadini, in particolare ai bambini e ai giovani. La severità della situazione pandemica dei Paesi centro-europei, ad esempio, che magari non hanno seguito il rigore dell'Italia, li ha visti costretti a misure drammatiche, con disagi importanti per i cittadini e per le attività produttive. La scelta di puntare sulla campagna vaccinale è stata una scelta vincente, vincente, come ci dicono i dati dei ricoveri e delle terapie intensive, e dobbiamo ringraziare la stragrande maggioranza dei cittadini che ha aderito alla campagna. La proroga dello stato di emergenza è quindi una scelta che viene fatta nell'interesse del Paese e della sicurezza di tutti. È errato pensare che lo sguardo reale sulla necessità di arginare determinati rischi che ancora possiamo correre alimenti le paure dei cittadini. Sono previsti tempi contingenti e certi che determinano questo importante passaggio di avvicinamento alla normalità. Abbiamo affrontato il problema delle scuole e degli atenei ben sapendo quanto la DAD abbia inciso non solo sulla qualità dell'offerta didattica, ma anche sullo stato d'animo di alunni e studenti, come pure di insegnanti e docenti che spesso hanno dovuto riadattare metodi di insegnamento, specialmente per i più piccoli. Non ci siamo dimenticati del disagio delle famiglie, disponendo, in un articolo del provvedimento, norme sui congedi parentali. La pandemia ha provocato uno sfilacciamento del tessuto sociale e ricostruirne la trama richiederà tempo e impegno da parte di tutti. È determinante, dopo una iniziale fase di grande incertezza, aver saputo e potuto, grazie alla ricerca, seguire gli sviluppi del quadro sanitario e delle mutazioni del virus, ma - voglio sottolinearlo dobbiamo un grande ringraziamento ai cittadini che, con grande senso di responsabilità, nonostante le paure, gli stravolgimenti della quotidianità e le limitazioni, hanno seguito le regole non sempre facili, rispettando il decalogo definito dalla scienza, ascoltando i virologi, coloro che dedicano la vita alla ricerca. Ora ci aspetta un tempo complesso, la ripresa dipenderà da molti fattori. Il nostro è un Paese capace di reagire. La mia Regione - lo ricordo spesso - nel 1976 è stata colpita da un terremoto devastante, ma i friulani si sono rimboccati le maniche come nel primo e nel secondo Dopoguerra per ricostruire i paesi e le vite dei singoli e delle comunità. Sono convinta, dunque, che saremo capaci tutti di riprenderci quella normalità che davamo per scontata e sulla quale anche questo provvedimento ci aiuta a riflettere per raggiungerla al più presto.

che sembra non avere fine. Da questi ultimi decreti che oggi discutiamo, che sono stati inseriti uno dentro l'altro come in una *matrioska*,

di mallevadori di una follia legislativa che ormai non conosce più limiti. Ormai le responsabilità sono solo politiche

tanta gente che ha contratto il Covid in questi due anni ha sicuramente un'immunizzazione più aggiornata rispetto a quella dei vaccini, e tuttavia non è esonerata dal dover fare dosi su dosi. Addirittura il personale sanitario sano viene estromesso estromesso e sospeso dal lavoro fino a quando non si vaccina, anche se immunizzato naturalmente. Siamo arrivati a questo delirio che ormai sembra non conoscere più limiti né confini, finalizzato esclusivamente alla vaccinazione. Addirittura vengono sanzionati i volontari che vanno a dare da mangiare ai senzatetto sotto i ponti,

che non hanno veramente alcun fondamento scientifico e su cui nessuno ha fornito spiegazioni, i genitori vengono costretti a vaccinare i figli pur senza

forniscono un'immunizzazione non aggiornata, e che, oltretutto, sui ragazzi e sui bambini è anche perfettamente inutile poiché questi riescono a superare il Covid senza conseguenze. Sapete benissimo che mancano studi sulle correlazioni con altre patologie; che mancano studi sull'efficacia - in termini di durata-effetto di questi prodotti. Sapete benissimo che mancano studi sugli effetti a medio-lungo termine e che, poiché avete definito vaccini questi farmaci sperimentali, sono previsti dalla normativa tre anni di monitoraggio addizionale che non sono stati per nulla attivati, perché siamo in farmacovigilanza passiva, e oltretutto i danni

al massimo ogni tre mesi. Non solo siamo in farmacovigilanza passiva e viene segnalato un effetto avverso su 100 almeno, ma oltretutto il *report* non viene fornito dal 12 ottobre:

se ci sono stati effetti avversi. Non sappiamo assolutamente nulla, però abbiamo i dati EudraVigilance su tutti i ventisette Paesi dell'Unione, che parlano di 38.983 decessi avvenuti in prossimità delle vaccinazioni e di 3.530.362 danneggiati. Questi sono i termini in cui dobbiamo parlare quando andiamo ad obbligare la gente a un trattamento sanitario a cui, se fossimo in a cui, se fossimo in un Paese normale, chiunque, facendo valere i suoi diritti umani, dovrebbe potersi sottrarre senza conseguenze sui propri diritti civili. Invece avete costretto la gente a scegliere tra diritti civili e diritti umani. *(Commenti)*. Adesso state pure colpendo i diritti politici delle persone, perché state limitando la possibilità delle persone vaccinate di essere rappresentate sia in Senato che alla Camera, escludendo tutti i parlamentari che non abbiano il super *green pass* che abbiano superato i cinquant'anni da qui al 15 giugno. Questo che senso ha sotto il profilo sanitario? Quale motivazione di natura sanitaria si cela dietro questa follia, visto e considerato che il tampone è l'unico strumento che viene effettivamente richiesto anche quando si tratta di situazioni particolari per poter attestare se una persona è contagiosa o meno, se è positiva o meno? Non dimentichiamo che avete consentito anche al personale sanitario, così come a tutti i lavoratori, anche positivo di saltare le quarantene se aveva la terza dose, perché - ebbene sì - con la terza dose ci si ammala - perché questo vaccino non immunizza - e si muore e si muore pure. Sono tutte fandonie quelle che andate a raccontare alterando i dati delle terapie intensive e dei ricoveri anche in in malattie infettive. Per quale motivo sono fesserie? Perché dalle stesse dichiarazioni dei medici e dei dirigenti ospedalieri vengono inseriti tra i non vaccinati tutti coloro che hanno superato i quattro mesi dall'ultima somministrazione di vaccino; tutti questi soggetti vengono considerati non vaccinati e inseriti in questo calderone. Pertanto, tutti i dati sono assolutamente sfasati. sfasati. Come potete permettervi di chiedere ai genitori di scegliere se far ammalare i figli per la loro mancanza di socialità, la loro mancanza di formazione e di scuola, o praticamente di esporli a un rischio biologico altissimo, su cui non fornite alcuna garanzia? Penso che a questo proposito ci siano veramente gli estremi per

Presidente, rappresentanti del Governo, credo che questa complicata legislatura che stiamo vivendo, con l'alternanza dei diversi Governi di cui abbiamo potuto fare esperienza in questi mesi, passerà alla storia anche per un obiettivo particolarmente qualificante che si è riusciti ad ottenere e che ha il nome di vaccinazione. Una vaccinazione che mai si era data prima in un momento storico senza che ci fosse stata una preparazione culturale. Ci siamo trovati davanti all'emergenza di una pandemia, e in tale emergenza abbiamo dovuto vivere il dramma delle morti, che adesso forse abbiamo anche dimenticato ma i cui numeri erano davvero pesanti,

del generale Figliuolo, che ha guidato queste operazioni e lo ha fatto - credo - con grande competenza e certamente anche con un piglio militare che non possiamo dimenticare.

di una patologia e di un'aggressione virale che ci ha lasciato nel mondo intero sorpresi, spiazzati, anche angosciati e rinchiusi in casa nei rispettivi *lockdown* lato, l'irruzione del vaccino come unico strumento, in quel momento, di risoluzione del problema: un mezzo di prevenzione che si innestava all'interno di una situazione ad elevata complessità e che ha cercato di creare, nella sensibilità di tutti noi, l'idea di vaccinarsi. Vaccinarsi fa bene: ricorderete tutti come, all'inizio di questa operazione, quella al vaccino sembrava quasi una rincorsa e sembrava quasi che l'azione del Governo fosse quella di rallentare, ordinare, classificare e stabilire le priorità, salvo poi, a un certo punto, innestare un'inversione di tendenza per cui era bene vaccinare tutti, sempre e comunque, fino agli *open day* della vaccinazione. Ma è stato proprio questo *pressing* positivo che ci ha permesso di emergere dalla pandemia, che non è ancora del tutto risolta, ma che comunque presenta presenta le condizioni o almeno le precondizioni per un ritorno alla normalità. Di questo stiamo parlando in questo momento: non tanto del *pressing* della vaccinazione che si è cercato di fare utilizzando tutte le possibili e immaginabili categorie: categorie: la persuasione, la convinzione e la spiegazione scientifica a quella dell'incentivazione (sappiamo di aziende che hanno addirittura promesso premi a chi si vaccinava), fino alla situazione opposta, che è quella della penalizzazione per chi non si vaccinava, quell'alzare sempre di più la quota di complessità della vita per chi si andava sottraendo al vaccino. Ora però questa sorta di emergenza richiede da parte di tutti noi lo studio di un piano inclinato per capire come ne veniamo fuori. Sappiamo che le situazioni più complesse sono, per esempio, quelle delle scuole: abbiamo creduto

Poi abbiamo scoperto che i bambini non erano affatto immuni dal rischio: ricordo all'inizio i primi casi che sembravano quasi orecchiare la sindrome di Kawasaki, che è una sindrome particolare, una patologia che colpisce i bambini, perché se ne coglievano le somiglianze e le differenze. Però certamente abbiamo visto bambini ammalarsi abbiamo visto quindi la necessità di estendere la vaccinazione anche a loro, ma soprattutto abbiamo tenuto conto di una cosa fondamentale: il bisogno di salute va sempre ottemperato all'interno di altri bisogni. Il diritto alla salute, previsto dall'articolo 32 della Costituzione, contempla la necessità, per esempio, che per i bambini si tenga conto del diritto all'istruzione, quindi del diritto a frequentare la scuola, e per tutti gli adulti del diritto-dovere al lavoro. Abbiamo vissuto l'esperienza dello *smart working*, abbiamo enfatizzato all'inizio come se fosse la soluzione e la panacea di tutti i mali, ma soprattutto abbiamo enfatizzato quello che riguardava la didattica a distanza. parlavamo della didattica a distanza come della soluzione ideale, anzi addirittura ne enfatizzavamo il valore per la spinta la digitalizzazione che stava offrendo.

oggi possiamo parlare della emersione dalla fase più drammatica e quindi del ritorno alla normalizzazione grazie a uno strumento: questo strumento resta, ancora oggi, la vaccinazione. Ancora oggi, in relazione alle terapie che ci permettono di intervenire per curare precocemente l'infezione che si stabilisce quando il virus attacca l'organismo, sussistono molte speranze e qualche dubbio, qualche perplessità. Sappiamo anche che, in questo momento, le persone che hanno ricevuto le famose tre dosi di vaccino e che comunque impattano, incontrano il virus possono cavarsela a volte con terapie che sono molto simili a quelle di una normale influenza; in qualche altro caso servono terapie più impegnative, come quelle con i monoclonali. con i monoclonali. Noi oggi stiamo discutendo come poter garantire alle persone quella vita normale, che include la possibilità di fare sport e di partecipare alle attività sportive,

ovunque la stessa ricaduta sul piano economico; non ha la stessa ricaduta sul piano, per esempio, della riapertura degli esercizi commerciali. Roma, da questo punto di vista, è una fonte continua e costante di esperienza di alberghi e di grazie a tutti che non solo ha ridotto le loro possibilità economiche, ma molte volte ne ha anche minato l'autostima, lo spirito di iniziativa, la voglia di rimettersi in gioco. In tutto questo influiscono non soltanto i costi emergenti, che sono in questo momento legati all'elettricità, alla luce e al gas, con tutto quello che ciò comporta, ma anche un'inflazione che sta rosicchiando condizioni economiche già provate dalla stessa pandemia. Ciò che noi chiediamo al Governo,

non riescono a vivere pienamente l'esperienza scolastica, nel caso dei ragazzi, e l'esperienza professionale, nel caso degli adulti. Abbiamo bisogno che in quei casi vi sia maggiore attenzione

più che un commento a questi due decreti-legge (perché sono due fusi in uno solo), che sono stati pensati un po' di tempo fa (era il 28 dicembre c'era una situazione epidemiologica ben diversa: era il picco massimo dei contagi, dei decessi e delle ospedalizzazioni), mi appresto a esprimere una sorta di auspicio nei confronti dei membri del Governo che sono qui presenti. Innanzitutto, visto che il quadro epidemiologico è cambiato (c'è stato un crollo, per fortuna vertiginoso, dei casi, quindi gli ospedali stanno cominciando a respirare e sono diminuite le terapie intensive), è bene che il Governo cominci a cambiare strategia.

i cittadini. Così lo diciamo una volta per tutte: è un obbligo surrettizio. Più obbligo questo dell'obbligo imposto per legge. Almeno siamo chiari, ce lo diciamo ed evitiamo le ipocrisie.

evitare il pugno di ferro, che magari li compatta tra loro e soprattutto li spaventa, ma cercare dialogo e confronto. Non ci stancheremo mai di dirlo: dialogo e confronto. Se i dati continuano a migliorare, come auspichiamo tutti quanti, se il virus diventa endemico e si va verso la fine dello stato di emergenza, bisogna cominciare a pensare di allentare le restrizioni; cominciare a pensare di archiviare il *green pass*, cominciando dal *super green pass*. Perché dico questo? Guardiamo a ciò che sta succedendo negli altri Paesi,

stop a mascherine e *green pass*: il Covid-19 non è più una malattia socialmente critica; in Francia revocheranno il *super green pass*. Allora, è plausibile che fra una settimana, invece, in Italia noi obblighiamo

Pensiamoci. Interroghiamoci su questo. I cittadini devono essere tutti uguali. Quindi, diamo la possibilità anche ai non vaccinati di lavorare e ai non vaccinati di venire in Parlamento a svolgere le proprie funzioni, che sono state attribuite loro dalla Costituzione. *(Applausi)*. Auspichiamo che il Governo intervenga in questa direzione, anche perché,

guardare i numeri reali e trarre le giuste conclusioni, perché non si possono continuare a considerare morti per Covid-19 coloro che non sono morti a causa del Covid-19, ma che sono morti per altri mali e avevano anche fatto un tampone risultato positivo, come aveva suggerito l'Organizzazione mondiale della sanità.

che i malati di Covid-19 vengono ristorati, a livello economico e a livello ospedaliero, in modo maggiore rispetto a tante altre situazioni.

è che se dessimo retta al CTS l'emergenza durerebbe quindici anni. È comprensibile perché, se non c'è più l'emergenza, viene meno anche il ruolo del CTS e, quindi, chi ne fa parte probabilmente non sarebbe più direttamente coinvolto in prima persona come lo è adesso. È umanamente comprensibile, ma attenzione: una cosa del genere alimenterebbe una cultura del sospetto fino a ieri ingiustificata. Qualcuno sarebbe legittimato a pensare che si vogliano abituare le persone alla sorveglianza e noi ci auguriamo che non sia questo l'obiettivo. La politica torni a essere protagonista, riprendendosi lo spazio che è stato lasciato in questa fase ai medici. La politica deve tornare a essere protagonista, usando buon senso e ragionevolezza.

Abbiamo sempre curato - giustamente, aggiungo io - assassini e clandestini perché sono persone, e ricordo queste parole scolpite. Se un cittadino italiano decide di non vaccinarsi, cosa facciamo? Non lo curiamo e lo lasciamo morire di fame? Scusate, ma da cristiani forse qualche domanda ce la dovremmo porre tutti.

Crisanti dice che oggi inseguire chi non vuole vaccinarsi non serve e non cambierebbe nulla. Francesco Vaia, direttore dello Spallanzani, ha detto di liberare le città dalla paura, restituendo la gioia di vivere. L'ossessione per il Covid sta generando insicurezza e aggressività. Stiamo attenti perché la gente ha voglia di ritornare alla normalità e non si può parlare di normalità associandola a libertà compresse.

e i vari decreti-legge afferenti sono stati emanati e l'attuale situazione generale. La situazione epidemiologica è sicuramente migliorata sia per il numero dei contagi sia per il progredire della della campagna vaccinale, che è riuscita a coinvolgere un numero sempre maggiore di soggetti che inizialmente l'avevano rifiutata aprioristicamente. Questa realtà è spesso il frutto di una campagna informativa che non riesce a toccare i tasti giusti o non è sufficientemente capillare nella sua realizzazione o, ancora, non riesce a trasmettere messaggi chiari e semplici, capaci di rimuovere remore o preconcetti legati - questi ultimi - spesso a soggezioni psicologiche o a retaggi culturali senza reale fondamento scientifico. il passare del tempo il muro di gomma si è allentato e sempre più cittadini aderiscono in modo responsabile alla campagna vaccinale, senza dimenticare il rispetto delle misure di protezione individuali e collettive, mentre le forme clinicamente gravi di Covid, quelle che richiedono ricovero ospedaliero o necessitano della terapia intensiva, hanno nei vaccini il loro punto insostituibile. insostituibile. La capacità di diffondersi e di contagiare del coronavirus, che è stata così alta per la variante Omicron, dipende in gran parte dal nostro senso di responsabilità; dal nostro senso civico di appartenenza a una collettività; dall'anteporre il rispetto della salute altrui, soprattutto per le persone fragili, anche rinunciando al giusto desiderio e alla voglia di riprendere a vivere, a rifare tanti gesti semplici di affettività e di condivisione di gioie e di dolori con i propri amici e i propri familiari. Ovviamente, però, se chiediamo ai cittadini sacrifici, restrizioni ed attenzioni, anche le istituzioni devono fare la propria parte. Tutto ciò deve essere realizzato in termini di programmazione, di scelte condivise, di corretto supporto e di adeguate capacità di risposta alle molteplici difficoltà e problematiche che colpiscono le varie categorie e le tante attività imprenditoriali e commerciali, senza dimenticare la necessità di un sempre costante e continuo coordinamento fra la cabina di regia centrale e le strutture regionali e territoriali. Non si può non rilevare che alcuni dei provvedimenti adottati e delle relative misure stabilite sono spesso il frutto di un compromesso politico tra le diverse posizioni di ciascuna forza politica. Tutti sappiamo che, per il bene del Paese, non si tratta di mettere una propria bandierina o di far prevalere una propria posizione, magari arrogante, senza condivisione, spesso legata a prospettive elettorali o alle sirene ammaliatrici dei sondaggi e degli *exit poll* del momento. Le scelte politiche - secondo me - devono partire da due punti fondamentali: da un lato, seguire le indicazioni scientifiche e le opportune valutazioni della situazione epidemiologica del momento, con le conseguenti previsioni del suo andamento successivo; dall'altro lato, verificare la corretta e capillare attuazione di quanto viene deciso. non si può prevedere l'utilizzo di mascherine FFP2 nelle istituzioni scolastiche, educative e universitarie - come d'altronde sono previste anche nel decreto-legge in esame, che stanzia a tal proposito ulteriori 5 milioni senza al tempo stesso verificarne la loro reale ed effettiva disponibilità in quelle strutture. Portando un altro esempio, occorre verificare che il prezzo calmierato dei test antigenici previsto per obbligo per le farmacie, per le strutture autorizzate e accreditate o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale sia realmente applicato secondo i protocolli stabiliti, evitando ulteriori aggravi economici per i tanti cittadini già in difficoltà. A tal proposito avevo presentato l'emendamento 14.0.6,

prossimi due anni in particolare) e monitorare i pazienti nel loro successivo decorso dopo la fase acuta del Covid dal punto di vista clinico, laboratoristico, cardiologico, pneumologico, ma anche psicologico.

sono previste a carico del Servizio sanitario nazionale, per due anni, alcune prestazioni come elettrocardiogramma, ecocardiogramma, spirometria e TAC torace per il *follow-up* di quei soggetti,

Avremmo avuto sicuramente un miglioramento di quanto si offre a cittadini per la tutela della loro salute. Occorrono scelte chiare, semplici, precise e lineari nella loro corretta applicazione, non ondivaghe o addirittura da sembrare concepite dalle menti di burocrati che vivono in una realtà lontana da quella che è la vita reale; o ancora - come in alcuni casi si verifica - provvedimenti adottati e modificati dopo alcune settimane, di cui i cittadini non riescono assolutamente a comprendere il significato. Vado a concludere, signor Presidente, ponendo l'accento su un altro punto di criticità. Ribadisco - secondo me - l'importanza di assicurare la piena attuazione delle misure per la riduzione delle liste di attesa, mai come ora estremamente lunghe; problema quest'ultimo indubbiamente già presente e quasi atavico su tutto il territorio nazionale, ma in particolare nelle Regioni meridionali. Occorrono necessariamente ulteriori interventi per garantire il recupero dell'arretrato causa pandemia, erogando prestazioni ambulatoriali di *screening* e di ricovero ospedaliero ordinario per patologie non Covid, che tuttora non risultano adeguatamente e tempestivamente prese in carico. Anche le opportune misure per contrastare queste criticità saranno l'espressione concreta di un effettivo ritorno alla normalità. Signor Presidente, il 4 febbraio è stata la Giornata mondiale della lotta contro il cancro: "*Close the care gap*", ovvero "eliminare la disparità delle cure", che è lo slogan scelto quest'anno. È necessario un piano di recupero per l'oncologia, per non avere, dopo la pandemia da Covid, accanto alle evidenti o quasi - oserei dire - inevitabili difficoltà economiche e sociali, una nuova emergenza sanitaria, una prossima epidemia di casi avanzati di tumore non più operabili o trattabili per i ritardi e le carenze accumulatisi negli ultimi due anni. Signor Presidente, vado a concludere. Il MoVimento 5 Stelle è rispettoso degli impegni assunti nei confronti dei cittadini e, pertanto, darà il suo voto favorevole al provvedimento in esame, pur con le piccole puntualizzazioni che ho voluto fare. Come ha ben spiegato e anche ribadito il nostro presidente Conte, vi è la necessità di un patto per i cittadini, di un'azione più incisiva per affrontare le diverse priorità urgenti, dal caro bollette, con risorse aggiuntive, agli interventi strutturali in sanità, senza dimenticare la sicurezza e la dignità del lavoro e le grandi sfide del PNRR e delle riforme. Queste sono solo alcune delle criticità e delle problematiche che ogni famiglia vive ogni giorno sulla propria pelle e a cui bisogna dare una risposta oggi, e non domani.

La Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto-legge, gli emendamenti 8.33 (testo 2), 8.0.5, 8.0.6,

Ma se chiediamo ai produttori e agli importatori di avere un prezzo calmierato nelle farmacie per le FFP2, non possiamo trovare nelle farmacie delle mascherine che non siano FFP2 vendute alle mamme e ai papà e che costano più di 75 centesimi e fino a qualche euro. euro. Non riusciamo a capire perché non ci sia la volontà di risolvere questo problema a due anni dall'inizio della pandemia. Quello in esame ci sembrava un emendamento di buon senso, perché si sa che le FFP2 per bambini non esistono, ma ci sono solo le FFP2 *small*. Quindi manteniamo questo emendamento e siamo felici che vengano coinvolti finalmente anche i produttori italiani che ci hanno dato una mano nell'emergenza quando le mascherine non c'erano. *(Applausi)*. È una cosa che probabilmente avrebbe dovuto essere fatta anni fa e non adesso.

perché non esistono tecnicamente, né da protocollo, mascherine ad uso bimbi. Quindi, cosa accade ai genitori, tra cui il sottoscritto?

impegni il Governo, che sta bandendo le gare e che già in questo decreto dovrà ottenere un rapporto di collaborazione diretta e di consultazione con i produttori italiani di mascherine che possono fare magazzino e programmazione nella filiera produttiva, ad inserire anche le mascherine FFP2 per bambini. Non stravolge il decreto, non stravolge l'impianto normativo e dà una mano a milioni di famiglie italiane con bambini che vanno alle elementari e in particolare alle medie. La FFP2 *small* a mia figlia non va bene:

di trovare una soluzione, con un ordine del giorno, magari firmato da tutte le forze politiche, che abbia una consistenza più importante come impegno al Governo, in modo tale che nelle prossime gare bandite dalla struttura commissariale siano inserite anche le mascherine per bambini. Questa è la richiesta e spero che il Governo possa considerarla, perché è una problematica quotidiana dei cittadini italiani. *(Applausi)*. Signor Presidente, visti il tema e l'importante attenzione che credo tutte le forze politiche vogliono dare a questo specifico argomento, proporrei, se possibile, chiedendo scusa ai colleghi perché abbiamo iniziato da poco, una breve pausa tecnica. *(Brusio)*.

Presidente, credo che la sospensione, se verrà accordata dall'Aula, sarà utile per confrontarci su questo tema.

Signor Presidente, per cercare di venire incontro all'esigenza di non far perdere tempo all'Aula e di non fare arrabbiare l'opposizione, chiediamo, come Gruppo Lega, se possibile - naturalmente dobbiamo essere tutti d'accordo - di accantonare momentaneamente questo emendamento

magari prima di allora riusciamo a risolvere questo problema.

Abbiamo una situazione che definire grottesca è dire poco. Abbiamo l'obbligo di mascherina FFP2 per i bambini, ma la mascherina FFP2 per i bambini non esiste. Non è una questione di dimensione, perché il bambino non è un essere umano in miniatura, ma ha una conformazione diversa. Un qualunque presidio medico non certificato per bambini non è adatto ai bambini; non è che, siccome è stato certificato per un adulto, lo facciamo piccolo e diventa per bambini. Ora, la domanda è questa: può il Parlamento italiano introdurre l'obbligo di una mascherina, se quella mascherina non esiste? La risposta dovrebbe essere lampante per tutti. Eppure non lo è. La risposta è no; eppure c'è l'obbligo di mascherina, anche se la mascherina non esiste. Davanti a una cosa tanto grottesca il Parlamento si dovrebbe ribellare. E infatti financo la maggioranza che sostiene il Governo dei migliori a un certo punto ha avuto un sussulto di dignità e un dubbio: possiamo andare avanti con l'obbligo di una mascherina che non esiste? Poi si sono radunati dieci minuti, si sono fatti due calcoli e hanno deciso che sì, si può stabilire l'obbligo di una mascherina che non esiste. il principio di realtà, cioè che quanto uno vede e vive è superiore a ciò che uno spera all'interno delle proprie ideologie, è alla base del comportamento umano e, a maggior ragione, alla base della politica occidentale. Ma noi ormai siamo arrivati all'esoterismo, che ha sostituito la scienza. Il Parlamento italiano pone un obbligo a cose che non esistono: obbligo di mascherina, ma la mascherina non esiste. È lo stesso che abbiamo visto con l'obbligo di mascherina all'aperto: è la più grande idiozia scientifica che sia mai esistita. *(Applausi)*. Il virus all'aperto e al sole muore, ma il Governo dei migliori, con il CTS dei migliorissimi, con gli scienziati prezzolati, ha deciso l'obbligo di mascherina all'aperto. Come il *green pass* per andarsi a comprare i calzini: se non hai l'autorizzazione del Governo, non puoi andare a comprare i calzini, non puoi andare a comprare un libro, non puoi andare a comprare il giocattolo del bambino, perché lo ha deciso il Governo dei migliori. Lo stesso che pone l'obbligo di una mascherina che non esiste. La verità è che questo Governo, che non esiste, è un Governo che ha sostituito la logica con l'ideologia e la scienza con l'esoterismo. Saremo sempre contrari a queste pagliacciate.

intervengo per fatto personale. Volevo dire al collega che io la dignità ce l'ho sempre, non solo in questo momento, fuori e dentro questo posto. Quindi moderi le parole, perché la dignità è una cosa seria e non si usa per propaganda politica.

di riconosciuto interesse unicamente in zona bianca (comprese quelle dinamiche e, quindi, in movimento). Abbiamo fatto fare il Festival di Sanremo al chiuso senza mascherina e abbiamo ascoltato il presidente Mattarella dire al Parlamento: rivendicate il vostro ruolo ed esprimetevi su qualcosa. una domanda ai colleghi. Se anche il Governo dovesse mantenere il parere contrario, questo Parlamento non è in grado nemmeno di esprimersi sulle manifestazioni che ci sono da centinaia di anni in questo Paese durante la guerra, con le epidemie e sotto invasione? Direi che non è il caso. Chiedo ai colleghi di tutti i Gruppi, a prescindere da altre posizioni ed emendamenti,

La curva è in fase discendente e credo che sia opportuno votare l'emendamento.

di avere, con il *green pass* base, quindi soltanto con il tampone, gli stessi diritti di chi vive nella Penisola. Il precedente emendamento ha una portata anche minore, perché questo estende estende la possibilità a tutti di utilizzare anche i trasporti aerei. Mi permetto di ricordare che per i trasporti aerei si è parlato in piena pandemia dei

Senatore Lorefice, l'approvazione dell'emendamento 2.1500/25 preclude in parte o assorbe il suo, per cui il suggerimento che le do è di sottoscrivere l'emendamento presentato

FFP2. Senatore Lorefice, credo che i due emendamenti impattino;

riconosce a coloro che sono sospesi dal servizio il riconoscimento dell'indennità alimentare, come per coloro che sono sospesi a causa di un procedimento penale. In altre parole, chiediamo che coloro che sono stati sospesi per l'imposizione di un trattamento sanitario godano almeno dello stesso trattamento di coloro che sono sospesi per un procedimento penale, cioè vengono trattati come i possibili

Signor Presidente, l'emendamento 9.3 riguardava la possibilità di effettuare i tamponi antigenici anche nelle parafarmacie. In questo momento ci sono file di cittadini davanti alle farmacie per effettuare i tamponi. È nostro dovere dare una risposta concreta, come è stato anche ricordato dal presidente Mattarella, seduta, nel precedente decreto-legge il Governo aveva già assunto l'impegno «a individuare le soluzioni più adeguate per assicurare la più ampia disponibilità per l'accesso dei cittadini alla fruizione di tamponi antigenici». non è stato realizzato nel decreto-legge. Quali interessi stiamo tutelando? Qualcuno dice quelli delle farmacie, perché in effetti con i tamponi si stanno fatturando importi elevati. Il margine di contribuzione per singolo tampone è in effetti generoso. Le farmacie però sono 20.000, mentre le parafarmacie sono 5.000 ed anche volendo, la riduzione del fatturato potrebbe essere pari al 18-20 per cento. Stiamo parlando veramente di poco. Il punto è che l'emendamento in questione era stato presentato nel precedente provvedimento dal collega Castaldi. Leggo dal resoconto di Commissione le parole del Governo: dalla relazione tecnica del Ministero della salute non si evince che tutte le parafarmacie dispongono di un meccanismo di accesso al sistema informativo di trasmissione dei dati ai servizi regionali. e delle finanze parlava solo di potenziali oneri derivanti da eventuali richieste di connessione al sistema della tessera sanitaria.

è stato ovviato all'unica richiesta del Governo, cioè la parte potenzialmente onerosa. L'aspetto grave è che il Governo non avrebbe dovuto non avrebbe dovuto esprimere in Commissione bilancio un parere contrario per assenza di relazione tecnica, in quanto la relazione tecnica c'era, era stato chiesto di verificarla e di andare oltre e controllare. La Commissione bilancio si deve esprimere solo

sul Covid, includendo anche tutti i laboratori di microbiologia e di biologia molecolare che non sono ancora inclusi e poi prevedere che siano accreditati certamente i laboratori con una certa esperienza di più di tre anni.

impegna il Governo: a valutare l'opportunità, nel rispetto dell'andamento della curva epidemiologica,

A questo punto, è forse meglio una sospensione di circa mezz'ora perché abbiamo la necessità di capire e chiarire. Ribadisco quello che ha detto il Presidente della Repubblica la settimana scorsa, quando ha rivendicato la centralità del Parlamento

a differire l'applicazione del decreto interministeriale che avrebbe ridotto le categorie tutelate. È stato un lavoro difficile e complesso in Commissione, un successo positivo, anche grazie al contributo di tutti gli altri Gruppi, atteso da molte persone che ricadono in queste categorie sfortunate. Dispiace rimarcare ancora una volta, purtroppo, che, dopo un lavoro intenso e fruttuoso in Commissione, al

tende a prevalere sulla volontà espressa dai rappresentanti del popolo. Abbiamo già detto più volte che crediamo che questa non sia una buona cosa e l'invito che faccio a tutti i Gruppi è quello di individuare soluzioni decisive e risolutive per evitare

collegato allo *smart working* che oggi viene rinnovato e prorogato per le categorie che hanno più bisogno in questo Paese. Grazie alla collega e grazie a tutti coloro che voteranno l'emendamento.

È iscritta a parlare la senatrice Binetti. Ne ha facoltà.

Passo al contenuto del mio intervento. In questi giorni si vive una distacco dalla realtà di ciò che avviene

che ci dicono che negli altri Paesi le restrizioni, gli obblighi e tutte le varie misure di contrasto alla pandemia vengono sospese, ridotte, se non annullate; in alcuni Paesi addirittura non le hanno mai avute.

La Danimarca le ha abolite, pur avendo un numero di contagi superiore a quello dell'Italia. La Svezia non ha mai avuto restrizioni. Negli Stati Uniti, anche gli Stati più rigorosi come quello di New York, si stanno abolendo pressoché tutte le restrizioni; molti altri Stati non le hanno mai introdotte. Il Texas ha abolito tutto dal marzo dell'anno scorso; il North Dakota e la Florida non hanno mai avuto delle restrizioni. Poi veniamo qui nel mondo irreale del Parlamento e del Governo italiano, che ne introduce di nuove, di più stringenti, di più irrazionali, di più inefficaci. Come ha ricordato questa mattina il senatore Zaffini nel suo intervento in discussione generale, l'Italia è uno dei Paesi con la più alta mortalità, pur essendo il Paese che ha le restrizioni più gravi; bisognerebbe porsi qualche domanda.

se si va a vedere la curva con le varie ondate di contagi e di decessi, naturalmente comparate alla popolazione, l'andamento è parallelo; a volte la curva della Svezia sale prima di quella dell'Italia, a volte dopo, ma l'andamento è lo stesso. La stessa cosa si osserva confrontando Stati degli Stati Uniti con politiche opposte come la California e la Florida, come il Nord e Sud Dakota, che hanno politiche opposte fra di loro, ma hanno lo stesso andamento.

Di fronte a queste misure, c'è veramente da chiedersi quale sia il senso. Noi abbiamo chiesto fin dall'inizio una serie di interventi al Governo. Il Governo è stato molto generoso nel limitare la possibilità di tutti gli italiani di svolgere una serie di attività; poi ci sono i non vaccinati che vengono sottoposti a una serie di restrizioni ulteriori, francamente ingiustificate in gran parte. Ma tutti gli italiani sono costretti, anche chi ha il famigerato *green pass*, a passare la giornata a tirar fuori il certificato e a farsi controllare per svolgere le attività della vita quotidiana (entrare in negozi, entrare in Parlamento, salire Parlamento, salire sui treni e sui mezzi di trasporto). Questo non è un privilegio, ma è un danno anche per loro: pensiamo a quante centinaia di migliaia di persone fanno questo tutto il giorno, e cioè controllare gli altri. Questo vale per le aziende e per le istituzioni pubbliche, con uno spreco di denaro e di tempo anche per chi ha tutte le certificazioni di questo mondo. Qual Qual è la ragione? Sono efficaci le misure adottate? No. Sono razionali? No. Sono giustificate da un fondamento scientifico? No. Già il comitato tecnico-scientifico ne ha fatte di tutti i colori, non ha azzeccato una previsione, ha detto tutto e il contrario di tutto. appreso poche sere fa addirittura che su parecchie decisioni è stato tenuto del tutto all'oscuro. Poi però il Governo ci viene a dire di aver seguito le indicazioni del comitato tecnico-scientifico: non è vero. Ci stiamo abituando a un Governo che mente sistematicamente al Parlamento. L'ha fatto il ministro Speranza, affermando di non avere operato presso l'Organizzazione mondiale della sanità per nascondere l'assenza scandalosa del piano pandemico in Italia; ci è venuto a raccontare che non era intervenuto e, poi, si è scoperto che era intervenuto. Questo si ripete: nella conferenza stampa sono stati mostrati dai numeri farlocchi e a poche ore di distanza il numero dei non vaccinati è aumentato di due milioni e mezzo. Succedono le cose più incredibili.

lo Stato non fa quello che dovrebbe. Noi abbiamo chiesto, praticamente da due anni, di lavorare per l'aerazione nelle scuole e finalmente in questo provvedimento, anche grazie a un nostro emendamento, nostro emendamento, se ne parla. Abbiamo chiesto il potenziamento dei mezzi di trasporto, ma non è stato fatto. Abbiamo chiesto degli interventi seri sulle terapie tempestive per tutte le altre malattie,

ha un tasso di mortalità più alto di quello degli altri Paesi, evidentemente si è sbagliato qualcosa. La vigile attesa, che in molti casi era inerte attesa, è costata dei morti; così com'è costato dei morti l'avere

Evidentemente, a lungo, le terapie non hanno potuto tenere conto di un fondamento della scienza medica da secoli, le autopsie, per capire cos'era successo nel corpo di coloro che erano deceduti. Non è stato fatto.

Fratelli d'Italia - che chiedeva una cosa molto europeista, e cioè che gli italiani avessero gli stessi diritti dei cittadini degli altri Paesi europei, ma addirittura extraeuropei. Va ricordato che chi ha fatto le due dosi da più di sei mesi, se è italiano ha perso il suo *green pass*, per cui non può più fare praticamente nulla, non può lavorare per moltissime categorie di persone, non può andare nei negozi, nei treni e così via; se però è straniero, per altri tre mesi può farlo. Ha senso questo? Dov'è la razionalità? Dov'è il profilo internazionale? Ci sono altre contraddizioni incredibili:

il sangue di una persona non vaccinata, ma quella stessa persona non può salire sul mio stesso treno, perché chissà cosa combina, dopo aver fatto il tampone e, quindi, avendo dimostrato che non è contagiosa? Ebbene, di fronte a questo noi votiamo contro il provvedimento in esame e chiediamo che il *green pass* sia abolito e si faccia ciò che serve agli italiani: le terapie, l'aerazione delle scuole, un'opera di informazione e non di propaganda, perché la propaganda - non è informazione - ha indotto scetticismo in moltissimi italiani, ottenendo il risultato opposto: gli italiani non ci stanno ad essere presi per stupidi e noi stiamo dalla loro parte.

Toninelli. Abbiamo apportato dei miglioramenti al provvedimento. Certamente questo è un decreto che è stato pensato in una fase completamente diversa.

di andare verso una riforma della sanità del nostro Paese. Abbiamo visto come siamo arrivati in affanno in pandemia. Poi, con i Governi Conte e Draghi, abbiamo ripreso la medicina territoriale; abbiamo reinvestito nella sanità pubblica. non siamo ancora alla fine della pandemia. Tutti vorrebbero l'endemia, che questo virus diventi una influenza. I dati ci dicono che non è ancora così. Certamente nella discussione c'è stata e c'è la cessazione dello stato di emergenza dal 31 marzo, ma io, ancora una volta, mi appello ai colleghi, mi appello alla politica. Noi abbiamo una funzione diversa, che non è quella

questo decreto nasceva a metà dicembre, in piena fase ascendente della pandemia. Quindi, serviva a dare un giro di vite e a dare maggiori tutele per quello che poi si è verificato, e cioè un picco impressionante dei contagi. Per fortuna, molte terapie intensive hanno avuto una crescita molto inferiore rispetto al passato, e questo anche grazie ai vaccini e dobbiamo ricordarlo. Come, però, c'è stata responsabilità da parte di gran parte del Parlamento, anche da parte del mio Gruppo, riconoscere la necessità di questo giro di vite, chiediamo che, con altrettanta correttezza e altrettanta responsabilità, anche l'altra parte del Parlamento riconosca che ora inizia una fase nuova. Inizia una fase in cui è necessario allentare certe misure restrittive, a cominciare dal *super* *green pass*, perché possiamo finalmente vedere la luce al di fuori del tunnel. Se i dati delle ultime settimane verranno confermati, potremo dire che finalmente la fase pandemica emergenziale sarà superata e potremo rientrare nella fase di gestione ordinaria. Questo è il nostro auspicio. Per quanto riguarda il decreto-legge, non posso fare altro che ricordare brevemente l'azione migliorativa che abbiamo svolto in Commissione,

messo su una bottiglia di latte, come il Ministro della pubblica amministrazione ha detto, ma è molto di più. Ricordo che ci ha salvato durante la pandemia dei trascorsi due anni disastrosi.

non consegno il mio intervento perché approfitto dell'occasione per salutare lei e i colleghi. Grazie a questo decreto-legge e a tanti altri sarò costretto a un lungo periodo di riposo forzato. Ne approfitterò per dedicarmi un po' al territorio, ma soprattutto ne approfitterò per disintossicarmi da queste Aule: un esercizio che, anche alla luce della futura composizione di quest'Aula e del taglio dei parlamentari, consiglio a tanti colleghi.

che non percepiranno un euro e saranno costretti a casa con le loro famiglie e i loro figli. *(Applausi)*. Sono preoccupato perché, in linea con i principi costituzionali, non stanno facendo altro che una consapevole e libera scelta.

Leggo la targa che la sovrasta: «Il 2 giugno 1946 per suffragio di popolo a presidio di pubbliche libertà e certezza di progresso civile fu proclamata la Repubblica Italiana». grazie a questa ricerca della libertà, soprattutto di scelta personale, in questa Aula in tanti anni, come tanti dei presenti ricorderanno, sono state combattute decine di battaglie, anche da parte di tante donne che adesso borbottano ai miei lati. la prima sul divorzio, ma anche quella sull'aborto. E si trattava di tante libertà che avevano al centro l'unica cosa importante per una democrazia completa: la libertà di scelta individuale senza creare danno ad alcuno. Ora ce ne sono tante altre di queste battaglie, cari colleghi, Presidente. Mentre noi oggi qui discutiamo di *green pass*, nei giorni scorsi si parlava della libertà degli uomini e delle donne di avere rapporti sessuali con chiunque, senza per questo essere bullizzati, stalkerizzati, picchiati o insultati in strada. Discutevamo della libertà, Presidente, di avere un mondo a colori, in cui uomini di diverse etnie, religioni e città di provenienza, potessero avere pari diritti e pari doveri. Discutevamo e discutiamo ancora addirittura della libertà di ammazzarci alla fine di un percorso di vita, di sofferenza e di malattia. L'unica libertà di cui non possiamo discutere è quella di rifiutare un vaccino americano che oggi, dati alla mano, non serve più a niente. *(Applausi)*.